Onorevoli Colleghi, giovedì 19 maggio è scomparso Marco Pannella, uno dei più grandi protagonisti della storia politica, sociale e civile del nostro Paese. *Leader* storico del movimento radicale, Giacinto Pannella, detto Marco, nasce a Teramo il 2 maggio 1930. La sua figura, complessa e vivace, è quella di un uomo autodefinitosi «radicale, socialista, liberale, federalista europeo, anticlericale, antimilitarista, non violento e gandhiano». È stato tutto questo e anche molto altro, ha rappresentato una voce critica, spesso in anticipo sui tempi, e un pungolo costante per le istituzioni. Nel 1955 è tra i fondatori - insieme a Ernesto Rossi, Leo Valiani ed Eugenio Scalfari - del Partito radicale dei Democratici e dei Liberali. Più volte parlamentare nazionale ed europeo, ha ricoperto anche la carica di consigliere comunale a Trieste, Catania, Napoli, Teramo, Roma e L'Aquila nonché di consigliere regionale del Lazio e dell'Abruzzo. Segretario del Partito radicale, Presidente del Partito radicale transnazionale e della lista Marco Pannella, nel 1977 fonda Radio Radicale, modello di servizio pubblico nella trasmissione dei lavori parlamentari, dei dibattiti politici e delle cronache giudiziarie. L'azione di Pannella si caratterizza per il costante ricorso ai metodi della lotta non violenta, modellati sull'insegnamento di Gandhi, al fine di affermare la legalità ossia - secondo le sue parole - «il diritto alla vita e la vita del diritto». È possibile richiamare soltanto alcuni tratti della sua vita politica così intensa, dedicata costantemente alla bandiera dei diritti civili e del garantismo. Pannella è uno dei principali promotori e protagonisti della campagna per l'introduzione del divorzio, culminata con la netta vittoria nel *referendum* abrogativo del maggio 1974. Due anni prima, anche grazie ad uno sciopero della fame, aveva contribuito ad ottenere la legalizzazione dell'obiezione di coscienza al servizio militare. A partire dalla fine degli anni Settanta promuove le iniziative del Partito radicale per l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, l'introduzione della disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza e la legalizzazione delle droghe leggere. All'inizio degli anni Ottanta, il suo impegno nella lotta contro la fame nel mondo risulta decisivo per l'approvazione della legge Piccoli, sui programmi di intervento nelle aree afflitte da emergenza endemica e alti tassi di mortalità. Dopo aver organizzato, insieme ad altre forze politiche, i *referendum* anti-caccia e anti-nucleari, Pannella, anche a seguito del clamore suscitato dalla vicenda dell'arresto e della condanna di Enzo Tortora, promuove, nell'ambito delle battaglie per la "giustizia giusta", il vittorioso *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati. Alla fine degli anni Ottanta è artefice della trasformazione del Partito radicale in movimento "transnazionale" e "transpartito", concentrato sugli obiettivi degli Stati Uniti d'Europa, della moratoria della pena di morte nel mondo e dell'affermazione universale dei diritti umani. Dal 2002, con la fondazione dell'Associazione Luca Coscioni, l'impegno si concentra sulla libertà di ricerca scientifica, la libertà di cura, la legalizzazione dell'eutanasia e del testamento biologico, il rifiuto dell'accanimento terapeutico. Tra le battaglie degli ultimi anni, ricordiamo quella per il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri italiane e per risolvere il problema del sovraffollamento degli istituti di pena. A tal fine, nel 2011, Pannella conduce con coraggio e determinazione il suo più lungo sciopero della fame, durato circa tre mesi. È di quel periodo il convegno «Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano», svoltosi, proprio con la partecipazione di Marco Pannella, il 28 e 29 luglio 2011 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, fortemente voluto dalla vice presidente del Senato Emma Bonino, che è presente in tribuna e che saluto.

A testimonianza dell'impegno disinteressato per la legalità e la democrazia, mi piace ricordare una sua affermazione, particolarmente significativa anche del tratto umano e dell'amore profondo e sincero per l'Italia: «Qualcuno mi ha chiesto quale sarebbe il primo provvedimento che prenderei se fossi eletto democraticamente Presidente. Ebbene, il primo provvedimento che prenderei sarebbe quello di dimettermi, perché, se il Paese mi eleggesse democraticamente, vorrebbe dire che non ha più bisogno di me». Gli attestati d'affetto di migliaia di cittadini in questi giorni hanno dimostrato il profondo legame che nella sua vita ha saputo instaurare con il Paese; anche chi non ha condiviso le sue battaglie e le sue posizioni politiche non ha mancato di riconoscere il sentimento di stima per un avversario che ha sempre fatto politica e mai cercato il potere. Nel rappresentare la commossa partecipazione del Senato della Repubblica al dolore dei compagni e della comunità politica radicale, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

Marco Pannella non ha mai fatto parte di questa Assemblea, ma non c'è dubbio che proprio al Senato sono legate due vicende molto importanti della sua battaglia politica,

per iniziativa e sensibilità del suo predecessore, l'amico Renato Schifani, Marco Pannella nel mese di luglio svolse a palazzo Giustiniani un importantissimo *meeting* sulle questioni della giustizia e fu in quella occasione il nostro collega Giorgio Napolitano, che onora quest'Assemblea, prese la parola per maturare quel messaggio di solidarietà e di condivisione

trasferito il senso di quell'intervento in un messaggio alla Camera e al Senato. Forse, signor Presidente, siamo stati interlocutori un po' distratti e a quel messaggio del Capo dello Stato non abbiamo prestato la dovuta attenzione. Oggi però c'è una situazione diversa. Al Ministero della giustizia c'è l'onorevole Orlando, esponente di tutt'altro schieramento politico rispetto al mio;

ho ascoltato, ho incrociato le parole di Marco Pannella. Forse non mi hanno convinto, ma come capita spesso con lui, qualche traccia c'è. Ritengo pertanto che, non necessariamente in memoria di Marco Pannella, come si è voluto fare ieri con l'iniziativa da me apprezzata del collega Manconi, si provi in questo fine legislatura ad abbattere quel muro costituzionale odioso che fu eretto nella scia

è preclusa e comunque è di fatto espulsa dalla Costituzione. Marco Pannella però è stato certamente tutto questo e anche molto di più. La sua più recente iniziativa qui in Senato fu l'estate scorsa. Vi partecipò l'amico sottosegretario Benedetto Della Vedova. Era un'iniziativa di ampio respiro internazionale, per lo Stato di diritto - come amava dire lui - contro la ragione di Stato. «contro la ragione di Stato» significava per Marco Pannella la classica contrapposizione dello Stato di diritto non alla ragion di Stato, che ha una storia precedente e che addirittura anticipa gli Stati moderni, ma allo Stato etico. Marco Pannella ha incrociato, talora confuso moltissime tradizioni politiche, ma dove c'era il cattivo odore dello Stato etico, Marco Pannella era Può essere significativo che, quando ha voluto tracciare un bilancio di se stesso e della sua esperienza politica - eravamo nel settembre 2014 fece un convegno bellissimo e scelse come suo riferimento Benedetto Croce, che significa lo Stato di diritto. Benedetto Croce in Abruzzo significava per Marco Pannella

Marco Pannella ha sempre avuto un profondo rispetto e affetto per la tradizione della destra storica, che poi veniva, colleghi, dal centro-sinistra di Cavour e Rattazzi.

Quello non può che essere, amici che venite dal PC, anticomunista perché l'Italia non ha avuto Léon Blum, come la Francia, ma ha avuto Ignazio Silone

«Non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu possa esprimerla». Questa fase, attribuita a Voltaire, filosofo francese del 1700, ben si adatta allo stato d'animo che oggi, noi della Lega, abbiamo in occasione del ricordo di Marco Pannella, recentemente scomparso. Molte battaglie da lui condotte all'interno e all'esterno delle Aule parlamentari non le abbiamo condivise, né sostenute. Abbiamo dissentito pesantemente da lui tutte le volte che, a nostro avviso, trattava alcuni temi, soprattutto quelli etici, come l'aborto, in maniera troppo Al contempo, non possiamo non ricordare i temi politici che ci hanno visti vicini e per cui abbiamo conseguito dei successi con le battaglie referendarie del 1995, dal *referendum* a favore della privatizzazione della RAI, a quello dell'abrogazione della norma che impone la contribuzione sindacale automatica ai lavoratori, a quello per abrogare la norma sul soggiorno cautelare per gli imputati di reati di mafia. Riteniamo giusto ricordarlo come un combattente. È il suo tratto caratteristico. Era impegnato nella lotta contro la povertà e la fame nel mondo e l'affollamento carcerario, anche se in merito abbiamo avuto e proponevamo delle soluzioni radicalmente - non è un giorno di parole - diverse da questi: lui con un pericoloso lassismo, che lo portava addirittura a sostenere la liberalizzazione e depenalizzazione dell'uso delle droghe, noi con la volontà di costruire nuovi istituti penitenziari. Marco, comunque, è stato uno che ci ha messo sempre la faccia e il coraggio, a costo di rimetterci la vita con, a volte, irresponsabili scioperi della fame e della sete, senza ipocrisie o convenienze del caso, al contrario di molti politici che lo hanno esaltato in morte malgrado lo avessero detestato in vita. A questo gioco abbiamo preferito sottrarci e, come Gruppo Lega, sia alla Camera che al Senato non ci siamo accodati a questo rituale. Abbiamo preferito evitare patetiche sfilate ed esibizioni a favore di telecamere, di telecamere, ma riteniamo doveroso ricordare l'uomo per il suo lungo ed inossidabile impegno politico e per avere inciso con il suo operato in cinquant'anni di storia il nostro Paese. Io, con i suoi interventi a radio radicale, ho imparato

Uno che non avrebbe mai rinunciato a ciò che doveva dire e a fare ciò che doveva fare, al punto da mettere la sua vita in pericolo. Vita che è stata segnata da lunghi scioperi della fame e della sete. A volte diceva molto, moltissimo, soprattutto quando si metteva il bavaglio. Noi, come Lega, lo ricordiamo così. Dalla mie parti però si dice che

Il problema è legato al fatto che una marea di inchiostro è stata spesa in questi giorni su Pannella. Lo consideriamo forse un atto dovuto, ma non sempre con una

Signor Presidente, colleghi senatori, le radici della formazione politico-culturale di Marco Pannella ci conducono su un terreno originale e non consueto. Marco era un liberale, e la contaminazione del suo liberalismo originario con motivi propri della destra azionista lo portò da un lato ad apprezzare il contributo dato dalla destra storica alla nascita del Paese e, dall'altro, in contraddizione apparente con questa sensibilità, a sviluppare una visione più liberista che crociana in ambito economico. Non si comprenderebbe Pannella, però, senza considerare l'influenza della nuova sinistra americana sul modo di fare politica prima ancora che sul terreno ideale. Provengono da Oltreoceano la non violenza, l'utilizzo del corpo come strumento di comunicazione e di lotta politica, la predilezione per azioni minoritarie che potessero conquistare la maggioranza agendo fuori dal palazzo e, anzi, in opposizione ad esso. Il Partito Radicale di Pannella, a differenza di quello di Pannunzio, Scalfari e di quelli che con loro andavano la sera in via Veneto, fu un fenomeno *post* sessantottino. Direi che fu il liberalismo possibile dopo quella stagione che, soprattutto in ambito giovanile, sconvolse il mondo. Fu il Sessantotto liberale e libertario che non involse in gruppetti settari e iperideologici. «Tu sei un rivoluzionario» scriveva Pannella ad Andrea Valcarenghi nella prefazione di «Underground a pugno chiuso», «Io amo invece gli obiettori, i fuorilegge del matrimonio, i capelloni sottoproletari anfetaminizzati, i cecoslovacchi della primavera, i nonviolenti, i libertari, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, i borghesi come me, la gente con il suo intelligente qualunquismo e la sua triste disperazione. Amo speranze antiche, come la donna e l'uomo; ideali politici vecchi quanto il secolo dei lumi, la rivoluzione borghese, i canti anarchici e il pensiero della Destra storica».

Il mio stesso percorso ne è una testimonianza. Studiavo in un liceo che ospitava tutte le formazioni dell'estrema sinistra, la Federazione giovanile comunista-italiana e un solo fascista. Quel gruppetto di radicali era un'ancora di salvezza per chi voleva sfuggire alle droghe delle ideologie novecentesche. Anche quando poi si prendeva distacco da quell'esperienza, come a me accadde a 22 anni dopo essere stato vicesegretario nazionale proprio di Marco, essa restava un punto di riferimento, prezioso pure per concepire idee differenti e a volte addirittura antitetiche o antagoniste. Oggi di luoghi di formazione, in fondo gratuiti e generosi, come quello che fu il Partito Radicale di Pannella, non ne esistono più. E questa è una perdita secca che condiziona la qualità della classe politica e quindi la ricchezza stessa della Nazione. Fu quello il periodo d'oro del Partito Radicale e del suo *leader*. Negli anni della cosiddetta Prima Repubblica le sue battaglie e lo strumento del *referendum*, del quale in seguito si sarebbe abusato, sconvolsero un sistema politico allora sclerotizzato intorno al bipartitismo imperfetto interpretato da due partiti-chiesa. Quando, nel 1976, i radicali entrarono in Parlamento, essi furono la prima formazione veramente nuova a riuscirci. Le grandi vittorie, dal divorzio fino alla battaglia su Enzo Tortora, appartengono tutte a questo periodo storico. Non è difficile comprendere perché, con l'inaugurarsi della cosiddetta seconda Repubblica, la vicenda politica e umana di Pannella, pur continuando a interpretare una testimonianza in alcuni casi al limite dell'eroismo, perde peso e incidenza politica. Il problema è che quella dinamica bipolare che nel corso della prima fase della Repubblica Pannella era riuscito a imporre sulle sue battaglie, tagliando trasversalmente la politica ufficiale e spiazzandola, battendosi per una legittimazione reciproca e generale che lo portò ad essere il primo *leader* a prendere parte a un congresso del Movimento Sociale Italiano di Almirante, e contrastando fino in fondo qualsiasi tipo di reato di opinione, a partire dal 1994 diventa la regola di funzionamento del sistema. In qualche modo, il bipolarismo si secolarizza. E la stessa cultura dei diritti civili cessa progressivamente di identificarsi con la difesa di una minoranza per diventare cultura di massa.

il quale, nell'intervento preparato per un Congresso radicale e letto postumo dopo il suo brutale assassinio a Ostia, rivolgendosi a Marco e a Gianfranco Spadaccia (che ha onorato le Aule del del Senato e che vedo oggi in tribuna e saluto), li implorava di restare irriconoscibili, per evitare che i diritti civili diventassero l'ideologia ufficiale dell'edonismo di massa e, per quella via, si facessero conformismo. Pannella quel rischio non l'ha corso, ma non ha potuto evitare - e probabilmente non l'ha mai neanche voluto - che il Partito Radicale di massa, come aveva capito Augusto Del Noce, nascesse altrove. In questa fase dell'attività di Marco non mancano le intuizioni folgoranti, come la comprensione che la globalizzazione avrebbe spostato le frontiere della lotta politica e che l'Europa, al di fuori dell'orizzonte fissato da De Gasperi e Spinelli, avrebbe rischiato l'implosione. se si guarda alla vicenda del Partito Radicale transnazionale e al tentativo di riformare il diritto internazionale, ci si rende conto di come un uomo politico che fin lì si era rifiutato di concepire la politica come gestione dell'esistente per provare a determinare il possibile attraverso la politica, fosse finito un po' fuorigioco, immaginando la politica come creazione dell'impossibile. Per questo il suo percorso negli ultimi anni si avvicina a una dimensione più laicamente religiosa che immediatamente politica: il rapporto con il Dalai Lama e la stessa lettera scritta a Papa Francesco prima di morire ne sono testimonianza. Tuttavia, oltre il percorso esemplare, resta qualcosa di urgente su cui riflettere al di là dei tributi di maniera. Si tratta di qualcosa che unifica la prima e la seconda fase del Pannella politico: l'acribia e il rigore, da destra storica appunto, con cui ha sempre insistito per il rispetto delle regole. Da qui l'attenzione alla qualità della legislazione come presupposto dello Stato di diritto e nutrimento del garantismo; da qui, come già detto, l'avversione nei confronti della criminalizzazione di qualsiasi opinione e nei confronti di qualsiasi reato di opinione; da qui, infine, la comprensione che nelle moderne società politiche la pienezza del diritto all'informazione, l'accesso ai mezzi di comunicazione e la possibilità per tutti di esporre adeguatamente le proprie idee, sono essenziali affinché una democrazia possa dirsi effettivamente liberale senza correre il rischio di diventare mera sovrastruttura. Queste intuizioni, esposte in maniera a volte prolissa, insistita, provocatoria, ricorrendo a un lessico originale e disordinato, attingendo parole nuove da quel canestro di cui ha detto De Gregori, restano materia viva sulla quale, oltre il tempo delle commemorazioni e oltre le appartenenze ideali che in quest'Assemblea ci dividono, bisognerebbe riflettere per onorare la sua memoria,

è stato iscritto al PSI dal 1987 al 1992, craxiano come me in quel periodo. Ha militato in molti partiti: dal Partito Liberale alla Rosa nel Pugno, ma con unico filo conduttore il suo il suo modo di vestire, con i*jeans.* Io sono uno di quelli che ha portato un mazzo di garofani rossi

le sue lunghe riflessioni a «Radio Radicale», le sue battaglie civili. Mi diceva che io avevo come strumento di lavoro la penna, altri il *computer*; lui come strumento di lavoro aveva il *referendum*

digiuni: lo sciopero della fame, quello della sete. Si scherzava sulla sua acidosi metabolica che - diceva - lo stimolava a riflettere e a dare di più; la sua disobbedienza civile (si è fatto arrestare), i suoi *sit-in*. Mi faceva la battuta che io da sindaco di Aulla avevo fatto il Comune dedipietrizzato e lui si doveva descalfarizzare: lo riteneva un errore che aveva fatto negli anni È questo Marco Pannella: un vulcanico uomo politico che stiamo ricordando, ma nella maniera che lui non vorrebbe; lui vorrebbe che lo ricordassimo con praticità.

non spendendo parole: lui ha bisogno di questo. È importante che il collega Manconi gli abbia dedicato un disegno di legge di riforma costituzionale con il suo nome, ma c'è un atto qui che è suo; non porta il suo nome

per ricordarlo per la sua vulcanicità, ma anche per la sua lungimiranza. Credo pure che dobbiamo riparare ad un torto ed è per questo che come Gruppo,

giorni nostri. Partecipiamo ovviamente al dolore di tutti i compagni e gli amici che lo hanno perduto e che non hanno più

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il fatto di commemorare Marco Pannella non nasce per me solo da un sentimento di sentita stima, ma da un sincero riconoscimento umano e politico ad un riformatore cui tutti noi - onestamente - dobbiamo qualcosa. Chi lo ha ricordato pubblicamente negli ultimi giorni ha tracciato la figura di Pannella come uomo politico, come amico, come collega e alcuni hanno perfino ricordato aneddoti di battaglie comuni e confronti politici. Personalmente non l'ho mai conosciuto, eppure mi sento coinvolto e sinceramente emozionato nel ricordare la sua personalità, così eccentrica, sognatrice, tante volte provocatrice, tenace, ma sempre onesta e coerente. Negli ultimi giorni ho riflettuto molto sulle sue idee; ho ripercorso, nei ricordi da semplice cittadino, la sua coraggiosa vita politica. Un aspetto, però, ricorreva sempre nella mia mente: il modo di interpretare la democrazia, quella diretta, nel senso più nobile ed autentico del termine. Con lui ha trionfato la visione più genuina della volontà popolare, capace di rappresentare il fondamento del nostro agire politico e sociale. Credo che, meglio di chiunque altro, nel corso della sua vita politica abbia saputo insegnarci l'importanza e il significato profondo della libertà, valore che spesso si apprezza solamente in termini materiali più che morali. Un altro saggio che ci ha lasciato ultimamente, ovvero Umberto Eco, definì Marco Pannella come colui che «ha insegnato agli italiani come si fa a diventare liberi, e soprattutto a meritarselo». Ha portato con sé, fino agli ultimi giorni, un grande ideale, che lui stesso definì un sogno: allargare la base sociale di partecipazione, anche tramite la via referendaria, alla vita politica e democratica, coinvolgendo attivamente i giovani, i cittadini, gli anticonformisti, coloro che non sempre si riconoscevano in un partito politico o in una ideologia ben definita. Sulle orme di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, ha intuito e denunciato tra i primi la crisi dello Stato nazionale, anche quando formalmente democratico, la sua inadeguatezza ad affrontare le grandi questioni del nostro tempo e i pericoli che l'illusione della sovranità assoluta dello Stato nazionale porta con sé. Pannella invocava la Patria europea contro l'Europa delle patrie e salutava il coraggio e la *leadership* politica del Dalai Lama nel chiedere, per il popolo tibetano, non l'indipendenza, ma l'autonomia, cioè la prospettiva federalista in grado di portare diritti e libertà anche per i cinesi e non solo per i tibetani. Indubbiamente è stato un grande uomo delle istituzioni democratiche e grande protagonista della vita politica del nostro Paese. Aveva un'idea esigente della politica, federale dell'Europa, laica dello Stato e rispettosa dei diritti individuali della persona. Le sue battaglie ne sono una testimonianza: basti pensare a quelle sul divorzio, sull'aborto, per i diritti LGBT e per l'ecologia (quando ancora un partito verde non c'era), per l'affermazione di politiche antiproibizioniste sulle droghe, contro la fame nel mondo o contro la disumanità delle carceri italiane, per una giustizia più giusta per il diritto delle persone a morire con dignità. Colleghi, diciamo la verità, oggi non parleremmo con tanta serenità di alcuni temi e problematiche se non ci fosse stato lui - con i suoi metodi e le sue provocazioni - ad aprirci gli occhi. Non oggi, ma ben trent'anni fa. Quale sia il giudizio che se ne voglia dare, Pannella ha contribuito a far diventare l'Italia un Paese più moderno, più civile e più libero. È questa la sua vera eredità, che va oltre le ideologie e le singole battaglie condotte nella sua lunga carriera. Concludendo, sbaglieremmo oggi a considerare questa vera e propria predicazione di Pannella come superata o utopistica. Pannella ci parlava - e il Partito Radicale continuerà a parlarci - di un'urgenza politica per l'oggi, della quale questo Parlamento e le nostre istituzioni dovrebbero farsi carico.

innanzitutto come senatori del Gruppo Misto e di Sinistra Italiana-SEL vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza al Partito Radicale e ai compagni di una vita, fino all'ultimo iscritto. Con Marco Pannella abbiamo condiviso molte battaglie: ogni volta che si è trattato di allargare i diritti civili e le libertà in questo Paese ci siamo trovati dalla stessa parte. Voglio qui ricordare non solo le battaglie che tutti ricordano, quelle per il divorzio e l'aborto, che hanno fatto fare all'Italia un salto di civiltà, ma anche quelle, magari più scomode, come la battaglia garantista, quelle per la difesa delle garanzie democratiche o quelle, per esempio, dei *referendum* sulla legge Reale o sulla legge 40, sul nucleare, sulla caccia, sui pesticidi e, soprattutto, le battaglie per i diritti dei carcerati. Cito quest'ultima questione non solo perché su questo fronte Pannella si è impegnato letteralmente fino all'ultimo giorno della sua vita, ma anche perché questa battaglia sacrosanta non è certamente ancora entrata a far parte del senso comune del senso comune degli italiani e del nostro Paese e certamente dell'agenda politica parlamentare. Se ne è parlato molte volte, si sono fatti annunci, ma le cose sono andate diversamente. Il solo modo per ricordare e onorare Marco è riprenderla e continuarla con la sua stessa determinazione. Sarebbe bene che i tantissimi che negli ultimi giorni hanno elogiato a gran voce le sue cause e la sua persona dessero ora seguito alle loro parole, rimettendo all'ordine del giorno quegli interventi di civiltà e umanità sulle carceri che sono stati sempre colpevolmente disattesi, firmando, per esempio, il disegno di legge il senatore Manconi ha presentato in queste ultime ore sull'Amnistia e indulto. Le battaglie di Marco Pannella sono state innumerevoli, troppe per citarle una per una, ma in queste campagne, che per decenni si sono susseguite una dopo l'altra e che potevano a volte apparire quasi casuali, c'era sempre una cifra comune: Pannella lottava per un'attuazione rigorosa della legalità costituzionale e dello Stato di diritto. Riteneva che fino a che i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione non fossero diventati tutti una realtà vissuta quotidianamente, la Costituzione non si sarebbe potuta definire compiuta né inverata. Anche dietro cause che parevano lontane da ciò, come quella per la liberalizzazione della *cannabis* o quella cui si era dedicato negli ultimi anni per il diritto alla conoscenza, era invece sempre presente l'idea di dover fare della nostra Costituzione e della legalità una realtà effettiva e viva. In queste battaglie Pannella ha messo in gioco tutto se stesso, il suo corpo e molte volte la sua salute, in quella lotta non violenta che ha insegnato a molti di noi a mettere in discussione il principio che il fine giustifica i mezzi perché molto spesso i mezzi, se sbagliati, mutano - eccome - il fine. Devo dire onestamente che quelle battaglie non le abbiamo condivise tutte, ma gli abbiamo sempre riconosciuto onestà, coerenza e assoluto disinteresse. Per questo anche quando difendevamo principi diversi e opposti - com'è capitato sul fronte dei diritti sindacali o su alcune scelte di politica economica o di intervento armato, per esempio, nell'ex Jugoslavia - non lo abbiamo mai visto come avversario. Pannella si proclamava ed era un liberal-democratico un liberal-democratico e, a differenza di molti altri che si definiscono liberali e democratici, lo era davvero. Per chi proviene da una cultura politica diversa era consolante e fecondo potersi confrontare

combattuta con la tenacia che gli era propria, abbiamo scoperto che questa vicinanza era condivisa da milioni di cittadini italiani. Credo che la vasta risonanza e la profonda emozione che la sua morte ha provocato in tutto il Paese riveli che nei confronti di Marco moltissime persone, moltissimi cittadini, provano un sentimento preciso e affettuoso: la gratitudine. Gli sono grati non solo perché in buona parte grazie all'impegno del Partito Radicale hanno oggi diritti che modificano e rendono migliore la qualità della loro vita, ma anche perché quelle battaglie, quelle campagne martellanti, che a volte parevano ossessive, hanno impercettibilmente modificato qualcosa di profondo nel senso comune del Paese e in loro stessi: quelle campagne hanno educato molti alla coscienza e alla consapevolezza dei loro diritti. Pannella aveva scelto di fare politica così: modificando il senso comune per incidere sulle scelte legislative, ma anche, in senso inverso, adoperando le leggi per modificare il senso comune e spostarlo sempre più avanti nel cammino di una società libera. Voleva essere, e in larghissima misura è riuscito ad essere, un uomo politico della strada e delle istituzioni allo stesso tempo. Marco Pannella è stato anche un pioniere della personalizzazione della personalizzazione della politica, nel senso che metteva in gioco la sua persona. Chiunque lo abbia conosciuto sa quanto fosse istrionico, plateale, spesso anche narcisista. Però non ha mai spinto la personalizzazione al punto di trasformare il suo partito, di cui era pure *leader* indiscusso, in "partito del capo", cioè in partito che avesse come bussola il successo personale del suo *leader* o del suo gruppo dirigente. La bussola resta sempre quella degli obiettivi, l'idea di società, di legalità, di Stato di diritto che i radicali avevano in mente. Del modello pannelliano, i partiti personalizzati di oggi hanno preso solo la scorza, mai l'essenza. Credo che Marco Pannella meriti da parte di tutti, di chi condivideva le sue battaglie come di chi le contrastava, un semplice riconoscimento: è stato uno dei pochi *leader* politici che ha saputo rendere questo Paese migliore.

a tutti coloro i quali hanno voluto credere nelle sue battaglie, a Rita Bernardini e alla mia *ex* vice presidente del Senato Emma Bonino, compagna con me di tante attività istituzionali programmate nella logica dei rapporti con l'Europa, nella logica della tutela della difesa dei diritti umani; una persona che ringrazio per essere qui, ringrazio per esserci, ringrazio per le sue battaglie, che siamo certi continuerà a fare con il sostegno di tutti coloro i quali hanno creduto nell'impegno di Emma e nell'impegno di Marco Pannella. Ho tanti ricordi di Marco e, quindi, non ho voluto preparare nulla di scritto, signor Presidente, perché quando si conoscono le persone, le lettere sono inutili e le parole a volte vanno pesate con il sentimento. Di Marco ricordo la forza delle sue battaglie, l'istinto di un sentimento convinto volto a realizzare quello che era il suo sogno: una giustizia giusta,

un lungo digiuno mi ha visto suo visitatore e suo ospite quando ero Presidente del Senato: siamo stati assieme a parlare dei problemi relativi alla giustizia, alla durata dei processi, allo stato di detenzione.

la politica è il forte sentimento del saper fare delle battaglie ed assumere delle scelte coraggiose (quali i suoi digiuni, che probabilmente lo hanno portato anche ad una lunga malattia), senza interessi senza nessun ritorno, ma soltanto con la condivisione di chi crede in quelle battaglie e nella forza di quelle battaglie. Marco era così. Ricordo tanti dibattiti telefonici su «Radio Radicale», il nostro caro amico Alessio Falconio, che ora dirige «Radio Radicale» e che prima lavorava qui in Senato per «Radio Radicale». C'è tutta una storia che mi ha visto seguire le sue battaglie assieme

Quando si è così e quando si assume questa identità forte, caratterialmente indistruttibile, non si può che lasciare un grande testamento, un testamento di coerenza, di forza, di trasparenza delle proprie battaglie, fino a soffrirne. Ecco, io penso che la politica debba riflettere su quello che ci lascia Marco e sulla vita di Marco Pannella. Mi auguro veramente di cuore che coloro i quali erediteranno il suo testimone - e ne sono certo, perché conosco le persone che mi stanno ascoltando - sapranno interpretare bene quello che è stato il suo percorso, perché noi, come Paese, abbiamo bisogno che gente come Marco Pannella possa portare avanti queste battaglie, possa portare avanti i temi etici della qualità della vita delle persone, della giustizia e dei diritti umani. Grazie, Marco Pannella.

in questo intervento non voglio fare una commemorazione ipocrita di Marco Pannella. Forse, per rendere omaggio veramente alla sua persona e ad uno dei grandi uomini della storia d'Italia, posso allora prendere spunto dalle sue stesse parole, che hanno definito il Movimento 5 Stelle come un fortunato incidente contro la partitocrazia. Proprio per questo, voglio raccontarvi che, quando il mio Gruppo mi ha chiesto di intervenire per fare questa commemorazione, ho avvertito un certo imbarazzo, perché si trattava per me di rendere omaggio ad una persona che, almeno inizialmente, non conoscevo. Poi ho riflettuto bene su ciò che è stato Marco Pannella ed ho realizzato che invece egli ha fatto parte anche della mia vita, come della

Posso ricordare, ad esempio, che Marco Pannella ha scritto molti articoli, ospitati anche sul *blog* di Beppe Grillo, tra il 2006 e il 2010, sui temi delle morti in carcere e sul proibizionismo; ci siamo rispettati e simpaticamente contestati più volte. «Agorà» fu la prima esperienza diffusa di Internet, nata nel 1993 per iniziativa proprio dei radicali. Nel 1993 le *e-mail* costavano 200 lire e con 50.000 lire si poteva avere un *account* sul sito «agora.it», un portale con tutti i siti Internet di politica e le prime *web* *chat*; un aspetto davvero pionieristico, che oggi sembrerebbe addirittura preistoria. Come tanti artisti, Marco Pannella purtroppo ci ha anche lasciato con tante battaglie ancora da combattere. Ad esempio ricordo l'uso della sua figura e di quella dei suoi compagni a livello mediatico. L'uso dei *media* per amplificare le questioni è stato, infatti, un tratto distintivo del suo modo di fare politica. Lo ricordo per come posso farlo, perché - ripeto - non voglio essere ipocrita. Quando mio padre, a metà degli anni Ottanta, annunciò a me, allora adolescente, che alle successive elezioni avrebbe votato per i radicali e quindi per Marco Pannella, io non capii quella scelta e anzi la considerai un un fatto ridicolo e scadente, proprio perché forse mio padre aveva rubato a me stesso quella parte di rabbia e di inquietudine che apparteneva a me adolescente, prendendosela lui. Pochi anni dopo, entrato entrato nell'età della prima maturità, ho invece compreso quella scelta che fece e penso che l'epoca fu giusto così. Come tutti i grandi artisti, Marco Pannella si è trovato da solo a combattere, perché aveva percepito, aveva aveva capito quello che gli altri non avevano probabilmente neanche visto; per questo molte delle sue battaglie sono ancora tutte da combattere; ovviamente, molte ne ha anche vinte: pensiamo ad esempio al alla sua rinuncia ai vitalizi, alla lotta per la liberalizzazione delle droghe leggere, alla sua lotta per il Tibet e alla sua amicizia con il Dalai Lama,

per quelli che sono stati i suoi tratti principali esso si è trasformato: la tribuna politica è diventata *talk-show*, il finanziamento pubblico ai partiti è diventato la legge Boccadutri, la partitocrazia è diventata lobbismo. Marco Pannella scrisse sul nostro *blog* che il petrolio è stato la benzina della corruzione e dei partiti e questa frase è probabilmente diventata una telefonata ad un compagno per annunciare l'approvazione di un emendamento. Io personalmente porterò con me il ricordo che ho fin da ragazzo di Marco Pannella: un uomo con i capelli bianchi che voleva migliorare il nostro Paese. Non so se lui abbia mai pronunciato il nostro *slogan* «mandiamoli tutti a casa», ma sono sicuro che almeno una volta nella sua vita lo ha pensato. Un saluto a Marco Pannella.

nell'ottobre del 1989 Marco Pannella, insieme ai colleghi Loredana De Petris, Valentini, Tocci e al sottoscritto, fu eletto nel Consiglio comunale di Roma,

che mise il Consiglio comunale di Roma in modo brutale di fronte a un problema reale e serio, quello di convivere con una persona malata di una malattia grave, incurabile e i cui

Marco Pannella ha poi sempre seguito le vicende del Consiglio nel quale era stato eletto fino all'autoscioglimento che abbiamo operato nel 1993.

Marco Pannella ha innovato molto la politica, anche nei toni, usando meccanismi anticonvenzionali, trasgressivi e clamorosi, che poi sono stati copiati, con una grande differenza: Marco Pannella utilizzava quegli strumenti per esaltare idee vere e problemi reali; spesso adesso questi meccanismi vengono usati per coprire il vuoto, lo zero pneumatico. Si occupava di cose pratiche; chiedeva denaro perché sapeva che bisognava far funzionare una macchina: dar vita a «Radio Radicale» e alimentarla. Sono certo che nessuno che ha dato una lira, un euro o un aiuto a Marco Pannella si è mai aspettato un qualsiasi tipo di gratitudine, diretta o indiretta, perché era una persona assolutamente libera, di testa e di pensiero. Il sistema giudiziario italiano è un servizio per il Paese che non funziona bene:

avrebbe cercato di dare una scossa. Non sono sicuro che avrebbe risolto i problemi; forse in alcuni casi li avrebbe creati, però penso che avrebbe messo una carica che forse al Paese sarebbe stata utile. Infine, penso sia stato un vero peccato che non sia stato nominato senatore a vita; lo avrebbe meritato perché certamente ha contributo a a fare dell'Italia un Paese più libero, aperto e tollerante. *(Applausi).* Sicuramente lo avrebbe meritato e sicuramente da questi banchi avrebbe rappresentato uno stimolo per il Senato a lavorare di più e meglio a favore dei cittadini. Penso che dobbiamo omaggiarlo con rispetto. e dicendo che sento molto il suo richiamo a non essere né ipocriti né conformisti nel parlare di Marco Pannella e della sua straordinaria personalità. Pannella ha fatto politica tutta la vita conducendo le sue battaglie sui diritti in solitario e con i suoi amici radicali. Sapeva scegliere gli obiettivi e, con la sua nave corsara, partiva all'attacco senza curarsi di maggioranze parlamentari e senza farsi condizionare da convenzioni sociali. Ha fatto lotta politica nel diritto e con il diritto. Ho condiviso molti dei contenuti delle sue battaglie, partendo da un punto diverso: ho sempre creduto nella Repubblica dei partiti, previsti dalla nostra Costituzione, che Marco bollava in blocco come «partitocrazia», parola insieme giusta e ingiusta perché non distingue tra il bene e il male, tra le degenerazioni della politica e chi tiene fermo lo spirito costituzionale e repubblicano. Rispetto alle navi corsare, è chiaro che i grandi partiti popolari sono meno rapidi nelle decisioni, più impacciati nell'organizzazione interna e sanno che ai diritti si debbono accompagnare i doveri e sentono il peso della concreta

ma dal punto di vista democratico, i grandi partiti popolari sono rappresentativi, stabili e quindi necessari. Queste due realtà, da un lato la nave corsara del Partito Radicale, e dall'altro la grande forza rappresentativa del Partito Democratico, sono la ragione di fondo della diversa posizione di due forze che spesso hanno condiviso analisi e obiettivi, sino ad essere talvolta presenti nelle stesse liste nelle elezioni politiche, come per esempio Emma, eletta nel 2008 al Senato come graditissima amata capolista del Partito Democratico in Piemonte e poi Vice Presidente del Senato. Nonostante le differenze, anche profonde, che hanno sempre segnato distanze non personali ma solo politiche, voglio dir qui, ricordando Marco Pannella, che la sua funzione nell'Italia repubblicana è stata molto alta, rilevante, incisiva. Si può dire, sapendo di dire la verità, che Marco Pannella è stato in tante circostanze il sale della politica italiana. Ci ha provocato, ci ha tenuti svegli, ci ha incitato e ci ha messi davanti ai grandi problemi del mondo: dalla necessità di abolire la pena di morte all'urgenza di far cessare le mutilazioni genitali femminili. Altrettanto grande, rispetto alla loro limitata forza parlamentare, è stato il ruolo politico dei tanti militanti radicali che, assieme agli azionisti, ai repubblicani, ai socialdemocratici, ai verdi e ai liberali, tutti parte di piccoli o piccolissimi partiti, hanno irrorato di cultura politica la democrazia italiana; l'hanno fatta maturare e resa più moderna. Assieme a Pannella, da molti decenni i radicali ci ricordano che talvolta non serve avere il potere per darsi grandi obiettivi e, se si è bravi, per vincere. Marco Pannella è ricordato e rispettato come protagonista influente di grandi battaglie che hanno traghettato un'Italia sonnolenta nell'era della modernità. Battaglie sui diritti portate avanti da piccole minoranze e battaglie sui diritti fatte proprie da tutti gli italiani democratici. Possiamo infatti dire, senza paura di essere smentiti, che larga parte degli obiettivi che Pannella si è dato nella sua lunga vita di lotte civili, anche se in partenza promossi da pochi, alla fine sono stati condivisi da larghe maggioranze di cittadini, anche da molti che gli erano politicamente distanti. Così è stato certamente anche per me, che non sono mai stato radicale ma che, voglio ripeterlo, ho spesso condiviso gli intenti delle battaglie che Marco Pannella lanciava o delle quali si appropriava. Tra tutte ne voglio ricordare una, che mi pare in fondo particolarmente nobile, disinteressata e significativa: la sua crociata contro il sovraffollamento delle carceri italiane per il quale, nel 2013, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Negli ultimi due anni l'Italia, anche sorretta dal toccante messaggio al Parlamento del presidente Napolitano, ha fatto molto per cancellare quell'emergenza e per restituire dignità ad esseri umani chiusi l'uno sull'altro nelle celle delle nostre carceri. È per il grande lavoro del Governo e di tanti, bravissimi, operatori carcerari, che è drasticamente diminuita la popolazione dei detenuti ed è fortemente aumentato il numero degli ammessi a quelle misure alternative al carcere che producono meno recidive e più sicurezza. Sono così venute meno le ragioni della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo e all'Italia è stato restituito il rispetto della comunità internazionale. Il ministro Andrea Orlando, che oggi è qui ha detto che quel poco o molto che l'Italia ha potuto fare per rendere più umane le nostre carceri non sarebbe mai stato possibile senza la spinta di due persone: una è Papa Francesco e l'altra è Marco Pannella. Pannella, ne sono certo, avrebbe apprezzato questo leale e meritato riconoscimento da parte del Governo. Ma non avrebbe certo perso l'occasione per dirci, con la sua ben ben nota intransigenza, che il nostro lavoro sulle carceri non è finito e che non dobbiamo fermarci sino a quando non avremo pienamente rispettato il dettato costituzionale che impone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Nell'intransigenza della difesa dei diritti delle persone che nessuno mai difende c'è la radice non solo del carisma di cui Pannella ha goduto in tutta la sua vita, ma anche della larga e sincera commozione che ha accompagnato la sua malattia e la sua scomparsa. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge

è con sincera commozione che prendo la parola in quest'Assemblea per ricordare la figura di Marco Pannella. Non voglio che sfumino o passino le parole e gli accenti che si sono ascoltati, anche in quest'Assemblea, e anche nelle scorse settimane, in concomitanza con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Le parole sono molto importanti e vanno sorvegliate quando si ricorda un politico e un uomo pubblico.

Nella comunicazione politica dell'Italia degli anni Settanta, paludata e ancora ottocentesca, i suoi *slogan,* le sue invettive e le sue espressioni provocatorie costituirono un'indubbia innovazione nella comunicazione. Si potrebbe dire che allora si aprì la strada a strumenti oggi tanto utilizzati e persino abusati. Lo si potrebbe dire, ma si sbaglierebbe perché gli *slogan* di Pannella non servivano la banalità e non erano a supporto delle parole facili. Certo, Pannella ha condotto battaglie che in qualche modo si stavano affermando nella società e usato parole d'ordine che in qualche modo corrispondevano a domande sociali che si stavano consolidando, ma ha condotto anche battaglie che apparivano alla società italiana lunari e distanti. Al servizio di queste battaglie egli ha messo la sua capacità di comunicare,

non per ricercare il facile consenso, ma perfino per seminare inquietudine e porre delle domande, perché erano l'altra faccia di quelle torrenziali comunicazioni, di quei discorsi fatti di frasi parentetiche e incidentali di digressioni di cui non si riusciva, se non a volte con difficoltà, a seguire il filo, perché erano il contrario della banalizzazione, costituendo il tentativo di rendere la complessità del tempo che stavamo e stiamo attraversando. In molti hanno voluto mostrare il loro affetto e salutare Marco Pannella nella casa in via della Panetteria, dove io stesso mi sono recato, accompagnato da quattro detenuti del carcere romano di Rebibbia. È una bella consuetudine dei radicali quella di recarsi in visita negli istituti penitenziari durante il triduo pasquale e nelle altre feste comandate. Quest'anno le condizioni di salute non hanno permesso a Pannella di lasciare la sua abitazione e così ho pensato di regalargli questa visita per dimostrargli la mia sincera gratitudine per l'impegno da sempre profuso dai radicali italiani e da lui stesso per i diritti dei detenuti. Il carcere - uso le sue parole - non può essere una «struttura di persecuzione sociale» per la soluzione di due problemi che non si sa altrimenti come affrontare: il consumo di droga e l'immigrazione clandestina.

(i riflettori che abbiamo provato ad accendere per migliorare le condizioni della detenzione e restituire alla pena il senso di umanità che la Costituzione gli assegna) lo dobbiamo anzitutto a lui e a Papa Francesco. Forse può riuscire singolare questo accostamento fra il vecchio *leader* radicale, libertario e anticlericale, e il Papa cattolico, gesuita, venuto da un Paese alla fine del mondo; ma c'è una parola, anzi un principio che li avvicina e che può avvicinare tanti di noi: la dignità dell'uomo. Questa fede tutta laica nella dignità dell'uomo, sostenuta da una fede altrettanto robusta nel diritto e nella libertà, ha costituito la stella polare dell'avventura politica e intellettuale di Marco Pannella; gli slogan utilizzati contro la demagogia e non a favore della stessa. Credo che non ci sia nulla di più vero nell'affermare questo, nel ricordare forse la sua ultima battaglia, quella, appunto, per le condizioni dei detenuti; quella di mettersi, in una società spaventata, dominata dagli imprenditori della paura, sostenuti da un'industria mediatica che fa spesso della paura il principale *business*, ecco, in questa temperie, mettersi dalla parte di Caino. Credo che proprio questo dimostri quella fede nella libertà e nella dignità dell'uomo, forse più di ogni altra battaglia. In un articolo che apparve anzitutto su un giornale spagnolo nel 1987, Leonardo Sciascia - che di Pannella fu amico e che fu vicino ai radicali fino al punto di accettare da essi la candidatura sia al Parlamento europeo che alla Camera - scrisse: «Pannella, e le non molte persone che pensano e sentono come lui (fra le quali mi onoro di stare) si trovano ad assolvere un compito ben gravoso e difficoltoso: ricordare agli immemori l'esistenza del diritto e rivendicare tale esistenza di fronte ai giochi di potere che appunto, nel vuoto del diritto, o nel suo stravolgimento, la politica italiana conduce». Non era un giudizio lusinghiero, per la politica italiana, mentre lo era certamente per Marco Pannella. È vero, Pannella ha dedicato la sua vita alle battaglie per lo Stato di diritto e la legalità, ed è vero anche che diffidava del potere, che spesso travolge o stravolge, con la sua componente innegabile di violenza, distorce, calpesta le regole del diritto e della democrazia. Non sarei sincero sino in fondo, non lo saremmo tutti, in quest'Aula, se affermassimo di condividere senz'altro l'idea, che Sciascia richiama e che tante volte Pannella ha ripetuto, a volte gridato, che la storia politica del nostro Paese sia stata gravata dal peso insopportabile della partitocrazia. Credo anche io, come Emanuele Macaluso - che ne ha parlato indicando una differenza di fondo rispetto al pensiero di Pannella che, forse, proprio la crisi dei partiti, che ha segnato questi ultimi anni, dimostri come da essa venga una maggiore debolezza, non una maggiore robustezza delle istituzioni della Repubblica. Eppure, nella sua denuncia e incapacità di cogliere quella denuncia, c'è un grande pezzo di irresponsabilità delle classi dirigenti che non seppero vedere la crisi di quel sistema e l'esigenze di reagire a quella crisi. Il mio racconto dell'Italia democratica e antifascista, nata dalla Resistenza, divergerebbe perciò in molti punti da quello offerto da Pannella, ma rimane salutare per la qualità della nostra democrazia e il suo mai sufficiente tasso di libertà quell'esercizio di diffidenza nei confronti del potere che Pannella non ha mai smesso di raccomandare. Uno studioso francese molto influente, Pierre Rosanvallon, ha parlato di controdemocrazia, a proposito di quelle forme di politica non convenzionale verso cui evolvono le esperienze democratiche dei Paesi occidentali. Credo che i radicali italiani e Marco Pannella si iscrivano pienamente in questo quadro. Non si tratta di un rigetto della politica o delle istituzioni. Al contrario, si tratta, per un verso, dell'eredità liberale di limitazione del potere attraverso il diritto, per altro verso, di forme di partecipazione democratica condotte su singole *issues*, definite in termini pragmatici e non ideologici, e spesso volte a richiamare i poteri elettivi al rispetto dei loro stessi impegni e della loro stessa legalità costituzionale. Mai la critica alla politica diventa sentimento anti-istituzionale. Nell'uno o nell'altro di questi registri si possono comprendere la gran parte delle battaglie che i radicali italiani hanno condotto, sotto la guida di Marco Pannella. Non solo quelle per il divorzio e l'aborto, durante la grande stagione dei diritti civili degli anni Settanta, per i quali credo che l'Italia debba essere grata a quest'uomo. Il *referendum* abrogativo della legge Fortuna-Baslini, che aveva introdotto il divorzio in Italia, si tenne il 12 e il 13 maggio 1974. Fu vinto dal fronte del «No» e, insieme alla sconfitta democristiana nelle successive elezioni regionali, determinò un profondo mutamento dello scenario politico e sociale nel Paese. La legge n. 194, sull'interruzione volontaria di gravidanza, fu approvata il 22 maggio del 1978, a distanza di circa tre anni dalla raccolta di firme promossa dai radicali per la depenalizzazione dell'aborto. L'Italia non avrebbe quella legge senza i radicali, anche se nel 1981 essi promossero un nuovo *referendum* per abolirne alcune parti, in favore di una completa depenalizzazione. Pannella e i radicali hanno però condotto la loro azione anche su altri terreni. Non posso non pensare, in particolare, alle campagne sui temi della giustizia: contro la legislazione emergenziale, per la responsabilità civile dei giudici, contro la carcerazione preventiva, per l'abolizione dell'ergastolo, per i diritti dei detenuti e per l'amnistia. È difficile negare che l'impegno di Marco Pannella abbia contribuito ad elevare l'attenzione e la sensibilità del Paese su tutti questi temi, anche quando più dibattuta poteva essere la posizione tenuta su ciascuno di essi. Allo stesso modo è difficile negare che in molti altri casi le sue intuizioni hanno anticipato un'evoluzione della politica e della società. Vorrei fare due esempi. Il primo riguarda la questione ambientale. È già nelle mozioni e negli interventi del congresso radicale del 1977 che si trova formulata una chiara linea ecologista, contro gli inquinamenti ambientali, le sofisticazioni alimentari, il consumo di suolo, per la promozione di leggi in difesa della natura e della salute. Lo stesso simbolo del «Sole che ride», utilizzato dai Verdi, fu loro ceduto dai radicali italiani. Oggi vi è una sensibilità ambientale molto più diffusa, sia fra i partiti politici che nella società, ma non v'è dubbio che l'ambiente e la sua tutela hanno smesso di essere considerati un lusso e sono diventati un parametro fondamentale nella produzione legislativa, anche grazie alla spinta radicale. L'altro esempio che voglio fare riguarda la proiezione transnazionale del Partito Radicale e il federalismo europeo. Non saprei contare le volte in cui ho sentito da Marco Pannella citare Ernesto Rossi, Altiero Spinelli o il Manifesto di Ventotene. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che Marco Pannella abbia trascorso più anni nel Parlamento di Strasburgo che in quello italiano, nell'arco di tempo che va dal 1979 al 2009, anni in cui gli Stati Uniti d'Europa sono stati per lui un sogno continuamente evocato e mai raggiunto. Di quell'impegno voglio ricordare in particolare un momento, assai significativo: l'istituzione, nel 1981, proprio per iniziativa di Altiero Spinelli, di una Commissione per gli Affari istituzionali, in seno al Parlamento europeo, incaricata di elaborare modifiche ai Trattati esistenti, allo scopo di promuovere la completa integrazione politica della Comunità europea. Vicepresidente di quella Commissione fa eletto il *leader* radicale. Anche in quel caso, credo si possa dire che Pannella era in anticipo sui tempi, e forse anche poco compreso: l'Atto unico europeo, che fu approvato nel dicembre del 1985, in Lussemburgo, non ridisegnava l'Unione secondo l'indirizzo del Parlamento di Strasburgo, ma si limitava a realizzare, entro il 31 dicembre 1992, il mercato interno. I temi politici rimanevano così elusi e l'Unione ne paga ancora oggi il prezzo. Mi accorgo che in queste mie parole sto forse nascondendo i tratti irruenti, istrionici, a volte irritanti, di una personalità ingombrante e, per tanti aspetti, fuori del comune. Nel rendere omaggio alle sue intuizioni e alle sue battaglie, sto forse lasciando in ombra uno stile politico che rappresentava sicuramente un'eccezione davvero singolare nel panorama italiano e, direi, europeo. Non voglio fare a Marco Pannella e ai radicali il torto di presentarli in abiti che non sono stati e che non potevano essere i loro. Non voglio perciò dimenticare i digiuni della fame e della sete, gli atti di disobbedienza civile, le provocazioni come quella di presentarsi imbavagliato in tv, per protesta contro la gestione dell'informazione da parte del servizio pubblico, o come la restituzione in piazza dei soldi del finanziamento pubblico ai partiti, con tanto di timbro impresso sulle banconote. Anche questa Assemblea, anche le istituzioni parlamentari della Repubblica e della Comunità europea sono state più volte «sfidate» - lo dico con il massimo del rispetto e della considerazione, ma anche della sincerità - dallo scandalo che Pannella e i radicali hanno saputo incarnare: penso alle battaglie ostruzionistiche, ma anche alle candidature controverse, promosse dai radicali. Ma corre anche l'obbligo di ricordare che il metodo non violento dei radicali e di Marco Pannella ha dato all'Italia pagine che rimangono scritte indelebilmente nella storia di questo Paese. Ha dato alla coscienza civile dell'Italia il caso di Enzo Tortora. Enzo Tortora fu arrestato per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico alle quattro del mattino del 17 giugno 1983, insieme a centinaia di altre persone, sulla base di dichiarazioni di pentiti rivelatesi in seguito del tutto false e infondate. Pannella ne sposò immediatamente la causa, e lo candidò al Parlamento europeo con un enorme rumore dell'opinione pubblica: come adesso, spinta spesso a condannare prima ancora di valutare e di comprendere. Dopo la condanna in primo grado, ad oltre due anni dall'arresto, Tortora venne eletto presidente del Partito Radicale, ben prima di essere definitivamente scagionato da ogni accusa. Bisogna dirlo: Pannella aveva visto giusto. E i radicali condussero un *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati, la cui onda lunga è arrivata sino in questo Parlamento, con la nuova disciplina approvata in materia lo scorso anno. Lo ricordavo in apertura di questo mio intervento e voglio ribadirlo: sui temi della giustizia, dei diritti, delle garanzie, sui tratti fondamentali di una civiltà giuridica liberale, la cultura radicale e Marco Pannella hanno offerto e continuano ad offrire un contributo imprescindibile. Il contributo si è prolungato anche fuori dei confini nazionali, con la battaglia per l'istituzione della Corte penale internazionale dell'Aia, e con la campagna contro la pena di morte nel mondo. Pezzi importanti non semplicemente della sensibilità, ma anche dell'ordinamento giuridico sovranazionale sono dunque legati all'impegno politico di Pannella e del Partito Radicale transnazionale da lui fondato. I fronti che Pannella ha aperto sono molti. Non possono stare tutti in un discorso; è davvero ammirevole come siano stati tutti in una vita soltanto. La campagna contro la fame nel mondo, quella per la legalizzazione delle droghe leggere, quella per l'obiezione di coscienza, le ultime battaglie sui temi della fecondazione artificiale e dell'eutanasia: mi limito a richiamarli in maniera così approssimativa per invitarvi a considerare come siano tutti temi sui quali la società non potrà che continuare a interrogarsi. Egregio Presidente, cari senatori, il 16 luglio 1974 - siamo all'indomani del *referendum* sul divorzio la prima pagina del «Corriere della Sera» ospita un dirompente articolo a firma di Pier Paolo Pasolini, con il titolo: «Apriamo un dibattito sul caso Pannella». Pannella stava conducendo in quelle settimane un lunghissimo digiuno per avere fra l'altro accesso ai programmi televisivi della RAI. E Pasolini prendeva di mira sia il clericalismo della Democrazia Cristiana di Fanfani, che il realismo politico del Partito Comunista, sordi alle istanze poste dal *leader* radicale. E all'uno e all'altro opponeva il candore di Pannella. Nell'incontrare l'ultima volta Pannella, a Pasqua di quest'anno, posso dire di continuare a non condividere la particolare durezza delle parole di Pasolini, ma, forse, di capire meglio cosa intendesse parlando del candore di Marco. Credo di averlo visto, quel candore. E anche se aprire un dibattito su Pannella era scomodo allora com'è scomodo oggi, credo che sia il modo migliore per ricordare un uomo al quale dobbiamo tante arrabbiature ma anche molta gratitudine. E credo sia giusto, proprio ora che lo salutiamo, provare ad aprire questo dibattito. Mi auguro allora che queste mie parole servano non a chiudere un capitolo della storia d'Italia, ma a svolgerne uno nuovo. Mi auguro infine che con questo stesso spirito di apertura al nuovo, di curiosità per i tempi che verranno, di disponibilità al confronto anche duro ma sempre leale fra le opinioni, di cui vivono le istituzioni parlamentari, sia possibile affrontare i passaggi sia politici che istituzionali

Signora Presidente, colleghi senatori, la proposta di legge che ci apprestiamo a votare va a colmare, direi finalmente, un colpevole vuoto normativo nella legislazione italiana. Mancava infatti un passaggio specifico e adeguato, sia nei contenuti, sia nelle procedure lasciate quasi *in toto* al lavoro degli enti locali e dei tanti volontari che lavorano in silenzio e con tenacia nel terzo settore. Per questo motivo e per lo spirito che la sostiene, sono particolarmente felice e orgoglioso di poter intervenire oggi in Questa legge passata alle cronache parlamentari e giornalistiche come provvedimento sul "dopo di noi", risulterà infatti importante e fondamentale per il nostro Paese. Tante sono le ragioni, come sapete, cari colleghi. Parlare del "dopo di noi" significa parlare di civiltà e dignità. Civiltà di un Paese moderno e dignità e autonomia delle famiglie e delle persone non autosufficienti con grave «diversa abilità». A molti di noi risulta spesso difficile comprendere il dramma autentico di chi si trova nelle situazioni che il testo vuole tutelare, ma non può essere più motivo di ritardi e causa di altri drammi. Per questo, lo sforzo e l'impegno come uomini delle istituzioni deve essere ancora maggiore, perché la politica deve essere attenzione a chi ha meno mezzi e possibilità degli altri. In caso contrario non può definirsi politica. Ma veniamo alla legge. Si tratta di un progetto che, come sapete, vuole garantire le prestazioni assistenziali ai diversamente abili in gravi condizioni che non hanno sostegno familiare. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spetterà poi individuare i criteri per regolamentare l'accesso ai benefici. Il legislatore individua negli enti locali, soprattutto i Comuni, i soggetti a cui è affidato il compito di assicurare l'assistenza. Speriamo che questa volta non si lascino soli come in passato, quando hanno dovuto gestire troppe emergenze senza chiari e dettagliati riferimenti legislativi. Questo è un punto importante che mi tocca personalmente. Prima di entrare in Parlamento, sono stato sindaco della mia città, Corato, in Puglia. I sindaci, non mi stancherò mai di ricordarlo, sono spesso i primi e a volte gli unici riferimenti dello Stato per i cittadini, coloro a cui per questioni delicatissime, come quelle del "dopo di noi", si rivolgono in prima battuta le famiglie. Bene. Già da sindaco, su una segnalazione, ahimè, drammatica e carica di speranze di un genitore, ho dovuto pensare ad un intervento che desse soluzioni a quella e ad altre famiglie. Grazie a un finanziamento nazionale e a un cofinanziamento comunale, siamo riusciti, e lo dico con orgoglio, pur in un momento di in un momento di tagli e ristrettezze finanziarie, ad inaugurare una struttura alloggio per diversamente abili in gravi condizioni, denominata proprio "dopo di noi", appartenente all'ente locale. Chi ha avuto un'esperienza come questa può comprendere gli impegni e, come dicevo, le speranze che si celano dietro tali progetti. Ma il fine giustifica i mezzi e gli sforzi: garantire un'adeguata assistenza ai soggetti diversamente abili privi dell'assistenza, materiale e spirituale, dei propri familiari. La realizzazione di quella struttura, diversi anni prima della discussione di questo provvedimento, costituisce oggi testimonianza non solo della sensibilità di quella amministrazione, ma direi esempio di ciò che va fatto da oggi in poi, senza abbandonare a loro stessi famiglie, figli, operatori socio sanitari, volontari ed enti locali. Lo ribadisco perché è in discussione, come dicevo poco fa, un principio di civiltà, dignità e solidarietà. Solidarietà istituzionale e umana nei confronti di chi deve continuare ad essere parte attiva delle nostre comunità. E non solo. È in discussione - lo ribadisco - il legittimo sostegno ai genitori, cui dare certezze e serenità,

su un'altra fase, denominata "durante noi". Si tratta di forme di coabitazione o "palestre di autonomia", anche per giovani che vogliano e possano intraprendere percorsi staccati dalla famiglia. Anche questi progetti richiedono, senza alcuna perplessità, adeguate forme di sostegno finanziario. In ragione di ciò, spiace individuare una nota dolente nel provvedimento in discussione oggi. Come Gruppo dei Conservatori e Riformisti condividiamo pienamente lo spirito del testo, ma facciamo notare che servono molte più risorse di quelle impegnate dal Governo per la sua attuazione. Affermiamo ciò a fronte del grande impegno richiesto alle comunità locali, sempre più prive di mezzi economici, strutture e personale. Il disegno di legge prevede infatti la costituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con diversa abilità grave, prive del sostegno familiare, con le seguenti dotazioni: 90 milioni di euro per il 2016, appena 38 milioni per il 2017 e 56 milioni annui dal 2018. Queste risorse vanno aumentate. Un altro aspetto di criticità che mi preme segnalare riguarda la metodologia di intervento, basata su provvedimenti parziali relativi solo ad alcuni aspetti della problematica. Tale approccio rischia di indebolire molto il ruolo di Regioni e Comuni nello sforzo di definire una programmazione coerente con i bisogni che il territorio manifesta.

Nonostante questi aspetti critici, ritengo però che nel complesso questa sia una buona legge, in grado di fornire le prime, sebbene non esaustive, risposte alle esigenze dei cittadini interessati, direttamente e non; risposte che - lo ripeto - il Parlamento può e deve continuare a dare. Signora Presidente, nonostante le tutele previste dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 162 del 1998, mancava un'iniziativa specifica a tutela delle persone con disabilità grave e per questo non autosufficienti, dopo la morte dei genitori o quando viene a mancare loro il sostegno familiare. Ci avevamo già provato nella scorsa legislatura, ma l'esame della proposta di legge non si era conclusa. Era stata fatta anche una petizione dalla deputata Argentin, che aveva raccolto quasi 89.000 firme. Finalmente in questa legislatura siamo riusciti ad unificare ben sei diverse proposte di legge in un unico testo, che ha l'obiettivo di evitare la sanitarizzazione dei casi più gravi, quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti, e di consentire loro di continuare a vivere nelle proprie case o in case famiglia

meglio individuata la platea dei beneficiari nelle persone con disabilità grave, così come definite dall'articolo 3 della legge n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Si è tenuto conto della necessità di far emergere con forza il superiore interesse delle persone con disabilità grave. Si è ribadita la necessità che le misure di assistenza avvengano attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e soprattutto nel

che disciplina i fondi speciali, ovvero nell'atto di costituzione del vincolo di destinazione siano indicati in carico al *trustee*, al fiduciario o al gestore, gli obblighi e le modalità di rendicontazione. L'altra modifica importante introdotta è stata quella di prevedere che in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* o stipulato i fondi speciali e costituito il vincolo di destinazione, i trasferimenti dei beni

Forse si poteva rivedere la questione dei *trust*, questa novità molto controversa, nella consapevolezza che non sono una soluzione per tutti, specialmente in un momento di larga diffusione della povertà. Forse si doveva approfondire la questione della disabilità intellettiva, che anche nei casi meno gravi è spesso associata ad altre patologie, come l'epilessia e l'autismo, quindi prevedere in tali casi la possibilità di usufruire di trattamenti simili a quelli contenuti nel presente disegno di legge. È anche vero però che nel Paese l'attesa era davvero tanta e se è vero (come è vero) che in Italia le persone colpite da disabilità grave e per questo non autosufficienti sono 2,6 milioni, il tempo è scaduto. rendere assolutamente un po' di serenità a quei familiari che vivono quotidianamente l'angosciante pensiero di cosa accadrà ai loro cari quando non ci saranno più, quando

un primo passo importante è stato fatto. Ora sarà importante continuare a tenere alta l'attenzione su quanto disposto dal disegno di legge; mi riferisco soprattutto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

le condizioni di vecchia e nuova povertà che, quando sono associate a situazioni di disabilità, sono insopportabili, esplosive e hanno un bisogno assoluto di tutta la nostra attenzione, di tutto il nostro impegno.

intervengo convintamente nel dibattito in corso su un disegno di legge che si attendeva da tempo e che riguarda il futuro delle persone afflitte da gravi disabilità. Sono quelle persone che, avendo una o più disabilità, eventualmente aggravate anche dall'età, non sono in grado di vivere una vita autonoma, che hanno bisogno di assistenza permanente e che hanno anche davanti a sé un futuro terribilmente incerto. Oggi queste persone vivono, se sono fortunate, con un parente prossimo (normalmente i genitori) che si preoccupa di fornire loro tale assistenza, spesso in totale solitudine. Detto per inciso, si tratta di un numero non indifferente di persone, in quanto su 3,2 milioni di disabili censiti in Italia ben 540.000 rientrano nella categoria dei disabili gravi, impossibilitati cioè a vivere una vita anche parzialmente autonoma. Non è certo il numero che ne fa una questione importante, perché l'assistenza a queste persone è la misura del livello di civiltà del nostro Paese. l'approvazione del provvedimento in esame sia un dovere per tutti noi. Ovviamente, come sempre, si poteva fare di più, a partire dai tempi, come diceva la senatrice

e i pazienti con gravi disabilità. Alla fine non vorremmo che il poco che si dà, in confronto alla spesa enorme che affrontano i Comuni

Pertanto, mi auguro che sia solo l'inizio di una revisione del sistema del *welfare* italiano in cui si riallochino risorse laddove sono più necessarie, soprattutto in aiuto alle famiglie. Abbiamo, infatti, il dovere di sollevare, per quanto si può, il peso che oggi grava quasi esclusivamente su di loro e contemporaneamente abbiamo l'obbligo civile di provare ad aumentare gli aiuti a domicilio, la possibilità di appoggiarci alle nuove tecnologie, di istituire residenze o case-famiglia che permettano la vita in un ambiente il più confortevole possibile e che eviti l'istituzionalizzazione dei disabili gravi nel momento in cui dovessero rimanere da soli. È per questo che uno degli aspetti più convincenti del disegno di legge è l'applicazione dell'istituto del *trust* anche alle situazioni di disabilità gravi, in cui i genitori potranno vincolare i loro beni, se ne hanno, ad un progetto di vita futura per la persona disabile quando loro non ci saranno più. Il provvedimento "dopo di noi" può rappresentare l'inizio di questo percorso e, soprattutto, una nuova speranza per tutte le famiglie che vivono nella disperazione e nel terrore del futuro

ulteriormente e convintamente, voterò a favore di questo provvedimento. Signora Presidente, ci troviamo a trattare questo tema dopo una lunga attesa e, in effetti, il tema è assai importante. È uno di quei quelli su cui si chiede al Parlamento di dare una risposta molto celere e concreta.

che piace al Governo e che la relatrice ha promosso in Commissione oppure il rischio reale è che si venga etichettati come coloro che non abbiano come interesse la soluzione dei problemi dei disabili.

Questo è un altro concetto che deve essere ben chiaro, perché troppo spesso si considera la disabilità come un problema arrivato in famiglia all'origine. Non è così: si può anche rimanere offesi durante la propria esistenza, e dunque è un problema che riguarda tutti. Come dicevo prima, a fronte di una disabilità, la prima questione che si affronta normalmente, come farebbe qualsiasi buon cristiano, è come dare cura e assistenza.

coloro che si prendono cura di una disabilità, piuttosto che di una malattia o di una difficoltà vissuta in famiglia. Un tema che riguarda un'altra legge, e non questo provvedimento, di cui abbiamo già sollecitato più volte la discussione in sede di Conferenza dei Capigruppo, e lo faremo ancora con estrema determinazione, perché dopo questo provvedimento si passi velocemente a dare risposta a quest'altra esigenza.

amorevoli delle cure familiari a coloro che hanno una situazione di difficoltà e la stanno vivendo. Non esistono situazioni prive di difetti. In queste ore, in questi giorni, scene raccapriccianti che vengono da Nuoro, con questi anziani che, ricoverati in case di riposo o in case di cura, sono malmenati da coloro che dovrebbero prendersene cura.

imperdonabile e sulla quale non può che esserci una forte reazione da parte della società civile.

Cosa accadrà dopo che la vita dei genitori o di chi è accanto alla persona disabile dovesse terminare? Chi si occuperà del disabile? Una soluzione prevista è quella dei *trust* non lascia totalmente privi da dubbi, in merito soprattutto alla possibilità che questo strumento possa essere a disposizione di tutti coloro che hanno il disagio da affrontare. il costo di un *trust*, in base a studi e analisi fatte, rischia di limitare forse al 5 per cento della popolazione disabile l'accesso a questo strumento. È uno strumento che appartiene a una legislazione non italiana, ma essenzialmente anglosassone,

Cito testualmente la sua risposta: «Il *trust* non è l'unico mezzo per attuare la legge. Inoltre, affermano che chi non potesse aderire a questa formula, può sempre fare riferimento ad altri fondi messi a disposizione dallo Stato per il mantenimento di queste persone con disabilità gravi».

limitato a una piccola parte della popolazione dei disabili. Se si parla delle altre risorse aggiuntive - bontà di Dio - in occasione di ogni manovra finanziaria assistiamo alla diminuzione delle risorse messe a disposizione per le disabilità gravi,

dando all'esterno una certezza di risoluzione dei problemi che è ben lontana dall'essere reale. Non intendo andare oltre, signora Presidente, rappresentando però fin da ora la mia difficoltà ad affrontare con

risorse non esistono. Il rischio reale diventa allora veramente l'istituzionalizzazione del portatore di *handicap,* in quanto la famiglia non è in grado di

altrimenti - ripeto - si vende per soluzione di un problema ciò che, nella realtà, si può tradurre come una limitazione alla libertà delle persone.

che hanno evidenziano con enfasi l'importanza del provvedimento, sia quanti, con grande trasparenza, lealtà e concretezza (penso all'ultimo intervento del senatore Candiani), hanno evidenziato anche i punti di criticità. Perché non dobbiamo nasconderci che possiamo fare di più, perché è ovvio ed evidente che le famiglie che affrontano condizioni di disabilità grave dei propri figli

assegnate dallo Stato ai Comuni pone sempre maggiori difficoltà. È ovvio che un fondo di 90 milioni di euro non può risolvere il problema

sottolineare in questo provvedimento come si sia guardato con particolare attenzione ai Livelli essenziali delle prestazioni. Questo perché lo attendiamo da tempo

del lavoro e del MEF di adottare entro sei mesi questi LEP almeno per quanto riguarda quanti sono colpiti da disabilità gravi mi pare un fatto particolarmente importante.

alla fine possa essere migliorato da questa Assemblea nella direzione che molti di noi auspicavano e rispetto alla quale in precedenza non era stato possibile andare. un ringraziamento sincero alla relatrice e alla Commissione competente per il lavoro svolto, anche perché si è tenuto conto di molte delle osservazioni che come Commissione sanità avevamo a suo tempo avanzato.

stante il livello avanzato di riflessione sulle modalità, sulle politiche, sulle strategie che possono essere messe in atto a livello territoriale, in una Nazione, per le persone con disabilità grave, forse molti di noi speravano di poter fare qualcosa di più avanzato. Non è stato possibile; siamo consapevoli delle grandi difficoltà di vario tipo (culturali, politiche, tecniche, economiche) che ci sono, e però, siccome poi

sia sottolineato nel momento in cui si darà attuazione, senza rischiare invece che sia privilegiata una parte che non è così chiaramente avanzata rispetto alle esigenze delle persone. Nel

che tutte le proposte devono vedere la partecipazione del disabile e della famiglia. Non c'è scritto che non lo si debba fare; l'importante è che chi darà attuazione a questa legge dia attuazione a quella semplice frase che, per fortuna, è stata inserita, deve essere il preminente interesse della persona disabile a guidare gli interventi. Questo basta, e speriamo sia sufficiente affinché il Ministero prima, le Regioni dopo, e gli enti che daranno vita ai progetti possano tenerne conto. secondo aspetto che voglio chiarire è il seguente: in tutti gli studi internazionali l'Italia è indicata come il Paese che, in Europa, soprattutto nelle politiche del *welfare* di tipo sociale, fa troppe erogazioni monetarie e offre pochi servizi.

ciò che verrà risparmiato potrà essere di nuovo versato nel Fondo per i servizi. Ciò che le persone con disabilità grave richiedono è infatti di aiutarli ad avere dei servizi adeguati alle loro esigenze, prima ancora che le erogazioni monetarie.

Luigi Santachiara, di 88 anni, si è tolto la vita impiccandosi al balcone della propria abitazione. In casa è stato trovato il corpo senza vita del figlio, Paolo Santachiara, di 51 anni, disabile dalla nascita e costretto sulla sedia a rotelle: egli è morto nel proprio letto, dopo che il padre gli ha tolto il respiratore e messo un nastro sulla bocca e sul naso. Il padre ha scritto in un biglietto, lasciato ai suoi familiari: «Scusatemi per il gesto folle». Scusatemi per il gesto folle... Qualcuno ce la fa e qualcuno non ce la fa: non ci sono "i migliori" e non ci sono "i peggiori", ma vanno aiutati tutti. tutti. È talmente grande il peso di un figlio gravemente disabile, che per reggere bisogna godere di ottima salute, soprattutto mentale, di buone risorse economiche, se possibile di molta fede, una buona dose di speranza e di tanta, tanta forza. Soprattutto forza e forza "sopra tutto". La forza di resistere alla disperazione, che si insinua nei modi più impensabili: il suo momento preferito è la notte, perché non si sa se ci si sveglierà. Mentre la stragrande maggioranza dei genitori pensa alle grane dell'indomani, all'amore della vita, all'ultima vacanza, al telefonino e a un mucchio di "vaccate" quotidiane, certe persone vengono assalite da una martellante ossessione: dopo, dopo di me, "dopo di noi" genitori, che sarà di lui, che sarà di lei o, addirittura, che sarà di loro? Ricordo infatti che qualcuno vive con più disabili a carico. I genitori disabili vedono il passare degli anni come l'angosciante allontanamento dalla meta, meglio, l'avvicinamento a problemi sempre maggiori, non alla soluzione di essi, come accade agli altri genitori. Ogni sera, spenta la luce, scalano un giorno dal tremendo conto alla rovescia, chiedendosi: e dopo, che ne sarà di lui? Lui che ha bisogno di mille accorgimenti personalizzati per funzionare, per avere un minimo di equilibrio, senza perdersi e persino senza morire. Chi davvero riuscirà a stargli vicino con le modalità e le tecniche acquisite, ma soprattutto con lo sconfinato amore di un padre e di una madre? Nessuno può dire adesso perché questi padri di famiglia siano arrivati a fare strage con un gesto estremo. Soltanto nel loro intimo riposano le segrete disperazioni e risposte che li hanno spinti fino a lì; e qui torna sempre il mantra, sempre quella terribile e inaccettabile frase che spesso sento anch'io e che diventa una preghiera quotidiana: "Signore, fallo vivere solo un minuto meno dei miei, un secondo, un giorno". Lui, genitore di disabile grave, non va in vacanza, non va al ristorante, non va con le amiche e con gli amici, se non quando avviene un vero miracolo sociale e organizzativo, magari grazie a qualche associazione benefattrice o al sacrificio di altri. Ogni cosa è vietata. Lui, la carne della sua carne, è sempre lì; lui ti aspetta, anche se non parla e anche se non te lo dice. Quanti sacrifici silenti, ogni normalità per lui è un lusso, una vera eccezione. Quante privazioni, quanti sacrifici compiuti da queste eroine; eroine, sì, perché sono le donne quelle che si sacrificano la maggior parte delle volte, anche se devo ammettere che conosco personalmente degli uomini, anch'essi dei veri eroi. Questo mondo di innocenti agli arresti domiciliari: questi sono i genitori. Sono degli innocenti agli arresti domiciliari. Questo mondo silenzioso di donne che ora mi dà voce e che vi urlerà pietà. Abbiate pietà e date dignità ai loro figli con una giusta legge. Abbiate pietà e date i diritti ai loro figli con una giusta legge. Abbiate pietà e date un futuro ai loro figli con una giusta legge. Abbiate pietà e date il dovuto ai loro figli con una giusta legge. Non concedete, non elargite, perché non c'è nulla da concedere, non c'è nulla da elargire. Bisogna solo riconoscere, riconoscere i loro diritti, quelli di essere creature umane, figlie di un Dio minore. Oggi sono solo i nostri figli, ma qui ha già accennato il senatore Candiani, domani potrebbero essere anche i vostri purtroppo. Non ve lo auguro questo, ma vorrei che voi ci pensaste a questa cosa. Potreste essere addirittura anche voi, perché disabili sicuramente si nasce, ma spessissimo disabili si diventa: basta un ictus, un arresto cardiaco, una pastiglietta in discoteca, un incidente automobilistico, una sciocchezza sportiva, un'aggressione subita, una malattia subdola e aggressiva. Fate una legge che non soddisfi le vostre supposizioni, il vostro pregiudizio e la vostra semplice pena passeggera. Ascoltate i nostri bisogni. Fate una legge che risolva i nostri problemi, non che acquieti le vostre coscienze. Fate una legge che risolva i problemi. Il *trust*, ad esempio, non è una priorità di nessuno. Nessuno di questi genitori. Il *trust* esiste già. Il *trust* per chi possiede denaro è già una possibilità e lo può fare anche oggi, non ha bisogno di questa leggiucola. Pensate non alla soluzione finanziaria, ma al disabile adulto. Lui è il figlio particolare, l'eterno bambino che ha bisogno di tutto, anche a 30, anche a 40 e pure a 60 anni. Anche a 70 anni; non che a 65 o a 66 anni diventi diverso. Qualcuno ha bisogno di essere imboccato, qualcuno sollevato, qualcuno curato, qualcuno semplicemente aiutato, ma tutte le diverse perfidie dell'*handicap*, soprattutto di quello psichico, sono accomunate da un'unica, granitica certezza: lui non può restare solo. Ecco cosa si intende per grave. È inutile che stiamo a correggere «disabile grave» o «disabile gravissimo». Dobbiamo distinguere i disabili mentali dai fisici. Lui non può restare solo. Ecco chi è il vero grave. Questi genitori vanno protetti e rassicurati da una legge che dia loro la certezza. Una legge che gli dia un conforto. Questo è il solo, unico compito di questa legge: farci invecchiare e farci morire in pace, serenamente, senza angoscia. Questo è un diritto nuovo che mi invento oggi: fateci morire in pace; visto che hanno compiuto tutta questa vita faticosa, almeno riconoscete loro il diritto di morire in pace. Quando poi succedono le disgrazie, quando poi qualcuno non ce la fa, chi osserva dal di fuori giudica; poteva suicidarsi solo lui? Poteva chiedere aiuto. Prima di giudicare, almeno provi a pensare. Sarà come restare fulminati da una rivelazione. Una rivelazione, direbbero i movimentisti di tutte le specie, indegna di un Paese civile. Questa Italia buonista, questa Italia nota per l'accoglienza, questa Italia così umana e sensibile,

Una rivelazione, direbbero i movimentisti di tutte le specie, indegna di un Paese civile. Questa Italia buonista, questa Italia nota per l'accoglienza, questa Italia così umana e sensibile, proprio questa Italia ha un'imperdonabile prerogativa: lascia soli i genitori dei disabili. Questa Italia che ha sperperato interi patrimoni pubblici nel modo più sporco e più bieco con la corruzione, l'evasione, la mafia, lascia soli i disabili e i loro genitori perché sono silenti. Ne volete degli esempi? Perché a questi genitori non è concesso un pensionamento anticipato? Lo abbiamo dato a milioni di italiani con le *baby* pensioni che abbiamo tutti sul groppone oggi, a a migliaia di politici e faccendieri fallimentari con trattamenti e buone uscite vergognose, e li abbiamo tutti sul groppone oggi. Questi genitori hanno un'aspettativa di vita di 17 anni in meno. Non lo dico io; lo dice un premio Nobel. Non un *blogger* qualsiasi che vivacchia di *click*. Con un'aspettativa di vita di 17 anni di meno non viene concesso un prepensionamento. Che cosa è questo se non un lavoro usurante? Perché a questi genitori non è riconosciuto a livello contributivo, assicurativo e sanitario tutto questo lavoro? Lavoro silente, lavoro invisibile, massacrante, usurante. I *caregiver* in Italia non sono ancora riconosciuti, mentre lo sono in tutta Europa. Candiani).* Di cosa hanno paura questi genitori? Che cosa temono davvero? Il 19 febbraio 2016 la polizia di Stato di Vercelli ha arrestato nel pomeriggio 18 persone per maltrattamenti a disabili; l'8 febbraio 2016, Grottaferrata: schiaffi, percosse, colpi col bastone della scopa, cibo fatto ingerire a forza, umiliazioni di ogni tipo, ma anche urla, insulti e minacce urlate a pieno volto a disabili. solo alcuni dei molteplici casi. Questa è cronaca; non sono sogni, non sono paure. Questa è cronaca. Dalla nascita, nelle scuole, dove se incontri un

l'articolo 17 di diritto alla formazione professionale; l'articolo 18 di diritto all'integrazione sportiva. Pur tuttavia, qualcuno lo dimentichiamo per andare in gita. Quando hanno 18 anni, gli è impedito di andare a scuola. Questo non lo sapete, ve lo dico io. A 18 anni li mandano a casa, non importa se hanno ottenuto o no il diploma. I nostri figli non possono finire le scuole; anche se sono in quarta, vengono lasciati a casa.

allo sport, come ho detto prima. Durante la fase adulta della disabilità, i genitori che accudiscono sono lasciati completamente soli e non parliamo del tabù più completo, della loro sessualità. In questa chiesa, oh, scusate, in questo Stato, è un tabù. Anche loro hanno diritto ad una sessualità. All'esterno c'è il *lovegiver*, qui se non è un «bunga bunga» o un «bingo bongo», non se ne può parlare. In queste famiglie quando va molto bene (perché l'eredità è ricca) il ricovero è in qualche struttura più o meno fidata e ben fatta, quando va male, è il *lager*. E delle differenze tra le Regioni? Voi sapete che, dopo le superiori, loro vanno a uno SFA, questi centri dove passano il pomeriggio. E gli SFA passano dall'essere gratis in alcune Regioni fino a costare 2.000 o 3.000 euro al mese in altre; nelle Regioni di mezzo si paga a metà, cioè metà lo paga il genitore e metà lo paga il Comune. E tutte queste differenze dove le mettiamo? Che altro vi serve per capire che queste persone hanno bisogno di uno Stato? Uno Stato che oggi non c'è ancora stato. Ogni soggetto che è un problema per la collettività dovrebbe in realtà essere una risorsa. Sì, pare incredibile, ma dovrebbe essere una risorsa; in primo luogo una risorsa d'amore e di carità, di spirito sociale e di condivisione di valori, valori non commerciali e non commerciabili. Conosco realtà che funzionano, da cui prendere spunto, ma sono poche. Sono piccole realtà che danno speranza e che non sono realtà all'ordine del giorno. Ne dovremo fare di passi avanti. C'è una mentalità da cambiare, un diritto da riconoscere, il diritto di esistere, di accedere, di percepire la vita stessa, di autodeterminarsi; il diritto di scegliere, di realizzarsi, anche nell'immobilità di sé o dei propri figli. «Scusatemi per il gesto folle», scrisse quel padre. Ma può un folle riconoscere e scusarsi della propria follia? No, miei cari, non era un folle, era un uomo che aveva consumato la propria speranza, la speranza che il figlio potesse avere il dovuto, il minimo dignitosamente dovuto. Ecco cos'è il nostro "dopo di noi". Eppure la nostra Costituzione, sotto la buffonata dell'assedio di Renzi, è chiara e palese. Articolo 30: «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». Si parla forse di età? No, si parla di Stato sociale, si parla di uno Stato che fa il genitore e che si cura dei propri figli. Allora smettiamo di riempirci la bocca con la parola "patria", quando continuiamo a dimenticare, se non a violare, la nostra Costituzione, mai applicata in molti e male applicata in altri dei suoi principi universalmente condivisibili. E non voglio proseguire con i due articoli successivi, ma non posso dimenticare l'articolo 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo Grazie, quello che questa legge dovrebbe applicare, se vogliamo davvero definirci uno Stato sociale. Queste sono le nostre paure. Quali sono le vostre proposte? Signora Presidente, quanti minuti ho ancora? PRESIDENTE. Ha ancora quattro minuti. n. 2232, "dopo di noi". Per molti di voi sono solo tre parole, io lo so che per molti di voi sono solo tre parole, tre parole che insieme non significano niente. Molti mi chiedono: che cos'è il "dopo di noi"?

Comunque, da stime effettuate nella relazione tecnica, si pensa che questa legge sia rivolta a 100.000-150.000 persone. Al comma 1 si evidenziano solo alcuni degli articoli della Convenzione ONU. Perché non è citata per intero? Perché solo alcuni articoli? Allora la citiamo tutta,

La Costituzione ci impone di togliere le barriere, non di metterle. Invece cosa facciamo qua? Mettiamo una barriera tra i disabili, dicendo che alcuni li aiutiamo

perché la differenza è stata sottratta per le detrazioni. In realtà stiamo quindi aiutando chi ha fatto degli investimenti, ma chi fa degli investimenti, chi fa un *trust*? Chi può,

Secondo un rapporto del CENSIS le persone con disabilità sono più di 4 milioni (questo è stato detto e lo lascio), ma vorrei dire che il 68,2 per cento dei contributi ricevuti dai disabili proviene dai parenti.

Si comincia quindi con una lunga vetrina di diritti, ma poi si mendicano *trust* e contratti assicurativi che portano solo sgravi fiscali a quanti hanno già una buona posizione economica. Peccato che chi compie questi gesti estremi, chi spera nello Stato, non possiede la casa, non ha altri redditi, e non chiede altro che di essere supportato nel lungo lavoro esistenziale da lui svolto. Non facciamo passare questo disegno di legge come rivoluzionario: esisteva già tutto. Tutto si compie alla Renzi, con botti e spettacoli,

intervento facendo un appello a tutti voi che in questo momento siete disabili; siete cioè disabili nel comprendere la gravità questo atto, vuoto di contenuti, tutto pieno di deleghe e di imprecisioni. Mi auguro che insieme lo si possa modificare in perché la disabilità è una questione di percezione: se si può fare una sola cosa, va bene se è necessario a qualcuno; adesso i genitori vi chiedono di fare una cosa bene

Presidente, gentili colleghe e colleghi, il presente disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 4 febbraio e poi dalla 11a Commissione del Senato, in sede referente, il 17 maggio scorso, reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno. Il provvedimento si inserisce all'interno delle materie riguardanti, da una parte, la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva dello Stato, e, dall'altra, la materia delle politiche sociali di competenza regionale. L'obiettivo, in estrema sintesi, è quello di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare, attraverso il principio della migliore collaborazione tra Stato e Regioni. È importante ricordare in questa sede la strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere il cui scopo principale è quello di mettere le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare

chiarisce i settori per azioni congiunte tra l'Unione e gli Stati membri. Accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione ma, soprattutto, salute e protezione sociale. Sono questi i punti chiave individuati a livello europeo come priorità per quegli 80 milioni di persone all'interno dell'Unione che presentano una disabilità da leggera a grave. È bene rammentare come la protezione sociale affronti questioni sociali diffuse sofferte dalle persone con disabilità quali la disuguaglianza di reddito, il rischio di povertà e l'esclusione sociale e come la salute garantisca che le persone con disabilità possano accedere in modo equo e sostenibile ai servizi sanitari e alle relative strutture. Per questo l'articolo 1 del disegno di legge, inserendosi all'interno di questo più ampio contesto generale di sviluppo a livello europeo, disciplina misure di assistenza, cura e protezione fondandosi sul rispetto del superiore interesse delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi

Quel «durante» esprime un concetto fondamentale, in quanto integra l'idea del "dopo di noi" arricchendola di contenuti e significati. Fondamentale, poi, laddove possibile, è il rispetto della volontà della persona, come richiamato nel medesimo articolo 1, ribadendo un principio che la legge pone al centro della propria struttura, ovvero il rispetto della volontà delle persone con disabilità o dei loro rappresentanti, affinché le relative decisioni vengano prese per il loro bene e con il loro supporto. L'articolo 2, ancora, in tema di prestazioni assistenziali e assistenza sanitaria, si fonda sulla collaborazione e sulla cooperazione tra Regioni ed enti locali,

che deve darci speranza perché non è un'elargizione, ma una risposta dovuta di una comunità civile e solidale come il nostro Paese è sempre stato. In questo Parlamento e in questo Governo l'attenzione c'è stata. Pensiamo soltanto alla legge di stabilità che ha stanziato 2 milioni di euro per le special Olympics

ma è il mondo della scuola che deve essere accogliente. Capisco che è sempre troppo poco, per tutto quello che serve e per un mondo che chiede ed ha tanto bisogno di attenzione. Ma questo abbiamo cominciato a farlo, e possiamo dire con gioia che

Signora Presidente, questo disegno di legge nasce con un nome: "Dopo di noi", quasi poetico. Sembra, per un momento, che realmente ci si voglia interessare alle problematiche dei cittadini, ma è solo un titolo, e come tale rimane, poiché il cuore del problema lo si vuole risolvere allargando la forbice tra Stato e privato, tra chi potrà essere accudito e chi no. Siamo coscienti del fatto che questo disegno di legge, l'ennesimo in questa legislatura, ha lo sgradevole olezzo di un atto scelto per alimentare clientelismo e interessi privati. È opportuno far notare che nel testo mancano i concetti base previsti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonostante essa sia stata timidamente menzionata nell'articolo 1. Le principali istanze, ribadite anche in modo estenuante durante le audizioni e che riproponiamo, sono: la possibilità per le persone con disabilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, e sul come, dove e con chi vivere; percorsi di transizione verso una reale deistituzionalizzazione, con azioni di progettazione indirizzate alla persona, finalizzate ad una vita adulta, alla partecipazione, all'inclusione sociale; misure di contrasto e di prevenzione della segregazione e dell'isolamento; misure e adozioni per l'accrescimento della consapevolezza; ma tutti questi riferimenti alla Convenzione ONU in questo disegno di legge mancano. Avremmo voluto che il disegno di legge fosse pienamente coerente con quanto previsto dalla

tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'uguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari». Mentre con questo provvedimento viene data alle famiglie un'unica possibilità di assistenza per i loro figli quando essi mancheranno, ovvero vedersi costretti a lasciare la loro eredità ai figli, ma non per gestirla come essi vogliono, ma per darla ad intermediari che la useranno per creare case-famiglia o addirittura trasformare i patrimoni e le case ereditati in case-famiglie. Questo

ma tutto è rimasto inascoltato e nel testo troviamo il *trust*, che la relatrice ha presentato e corretto con ben tre subemendamenti. L'emendamento della relatrice è stato scritto proprio per dare legittimità all'eventuale introduzione nel nostro ordinamento di questo istituto, senza però chiedere parere di merito alle Commissioni finanze e affari costituzionali, oltre alla Commissione giustizia. Risulta quindi un vuoto normativo non di poco conto. Questo - a nostro avviso - è estremamente grave; si vuole forzare il *trust*, dandone consistenza tramite un che ne introduca l'istituto, poiché appunto, non è presente nella normativa italiana. L'emendamento della relatrice oltre a prevedere la figura del *trust* come strumento giuridico da impiegare in favore delle persone con disabilità, introduce la figura del *trust* "auto dichiarato" ovvero il caso in cui fiduciario e fiduciante coincidono. In questo caso mancherebbe un un trasferimento di beni e sussisterebbe solo un vincolo di destinazione degli stessi. In parole povere, il proprietario di uno o più beni li separa dal resto del suo patrimonio e li destina per determinati scopi. La Cassazione ha fortemente criticato questa particolare figura di *trust* auto dichiarato, che non può assolutamente qualificarsi giuridicamente come tale. In pratica si sta definitivamente scegliendo di indirizzare le risorse per la tutela e la gestione della vita delle persone con disabilità verso l'iniziativa privata quasi come se lo Stato dovesse inesorabilmente arretrare, rinunciando al suo ruolo primario, rispetto alla tutela dei diritti inviolabili dei più deboli, lasciando che la risoluzione dei problemi di queste persone sia appannaggio di iniziative privatistiche, perseguendo gli interessi di pochi e non certo l'utilità sociale!

il contratto di affidamento fiduciario, denota una visione miope e di assoluta disparità sociale. Questa politica di trasferimento del sistema socio-sanitario dal pubblico al privato è stata fotografata dal Censis, che ha certificato come nel 2014 vi sia stato un aumento di un miliardo della della spesa sanitaria privata. Ricapitolando, la fase emendativa al Senato si è distinta dapprima per l'introduzione nel testo dell'istituto della fattispecie contrattuale atipica del contratto fiduciario, che ha fatto sorgere forti dubbi sui possibili impieghi in tale campo, dato che si tratta di un istituto giuridico che, per quanto astrattamente legittimo, nella prassi può dare origine a operazioni opache e non certo trasparenti. Sebbene sia ammissibile nel nostro ordinamento, in virtù di quanto disposto dell'articolo 1322 del codice civile, nella prassi tale viene talora impiegata come espediente giuridico che cela operazioni contrattuali talvolta simulate con cui dare origine a operazioni fittizie o artificiose al limite della legalità. In ultimo, è previsto l'impiego del contratto di affidamento fiduciario, altro istituto non proveniente dal diritto positivo, ma di origine dottrinaria. un contratto con il quale l'affidatario fiduciario (magari una fondazione) gestirà, secondo un programma, i beni nell'interesse del beneficiario persona disabile. Il problema non è tanto questa figura contrattuale, quanto capire perché il legislatore deve ricorrere in tale sede a tali strumenti giuridici, lasciati alla libera iniziativa privata, non codificati, per disciplinare un problema di carattere generale quale la vita e il futuro delle persone disabili. Sembra una forzatura e lo è. Non si comprendono, poi, quali siano i reali vantaggi per una famiglia derivanti dalla stipula di polizze assicurative, come previsto dall'articolo 5, poiché il risparmio è assolutamente esiguo. Il beneficio di questa misura per le famiglie è sovrastimato in ragione della detraibilità di imposta e il vantaggio che porta è realmente modesto. stato più in linea con le reali esigenze adottare un sistema analogo al regime tributario previsto per le forme pensionistiche complementari, così da gettare le fondamenta per dare concreta attuazione al progetto di vita individuale in modo parallelo e complementare alle risorse messe a disposizione dallo Stato.

ancora maggiore attenzione. Si tratta di una fascia di popolazione a cui - è un imperativo categorico - lo Stato deve dare assolutamente risposta.

noi" restituisce sicurezza e maggiori certezze a quegli straordinari, sì, quegli straordinari genitori dei ragazzi disabili gravi; alle famiglie che rivolgono a questi ragazzi la loro intera vita, dedicandogli la massima cura nella ricerca di un futuro, perché devono poter trovare Sino ad oggi questo passaggio del testimone ha visto le famiglie perlopiù sole. Oggi anche lo Stato vuole essere loro più vicino: uno Stato che ha il dovere costituzionale

Governo, colleghi carissimi, siamo di fronte ad un disegno di legge sul quale mi soffermerò brevemente proprio per illustrarne alcuni passaggi fondamentali. Si tratta di un provvedimento che, com'è stato detto già da molti di noi,

sostengono i propri figli nel momento in cui hanno una forma di disabilità che si concepisce anche nel rapporto con l'ambiente circostante.

contenuti importanti. Saranno sicuramente perfettibili, saranno soggetti al vaglio di un monitoraggio, ma certamente sono un passo che ci è stato chiesto e che noi siamo stati in grado di fare. fare. Ho sentito molto spesso citare la parola «*trust*» negli interventi di tanti nostri colleghi che

ovvero non limitarsi al solo *trust* come forma giuridica, perché i genitori potessero sentirsi tranquilli nel momento in cui venissero a mancare per i loro figli, ma anche durante la loro vita, nel momento in cui venissero a mancare le forze per sostenerli. Sono stati aggiunti fondi speciali e vincolati quei fondi aprendo a tutte quelle associazioni che si muovono prevalentemente nell'ambito del volontariato. Abbiamo risposto con coerenza ad una richiesta molto precisa e molto ben definita.

esso rimette gli enti locali e il Governo nella condizione di dover in qualche modo riconsiderare una serie di parametri.

la condizione funzionale differente rispetto a quella che chiamiamo "normalità" non potrà essere superata, ma potremo garantire dignità di vita a queste persone e farle diventare

oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare». Si tratta di un intervento normativo di estrema rilevanza sociale, perché, attraverso questo testo, abbiamo l'opportunità di incidere sulle vite di una categoria di cittadini, che da tempo necessita di maggiore attenzione e tutela. Il nostro non è un Paese in cui la vita sorride sempre, nemmeno per un cittadino giovane e in salute, ma è un Paese in cui, spesso, le categorie deboli, svantaggiate, impedite, sono abbandonate a se stesse, in una logica quasi darwiniana di selezione della specie: solo chi è abbastanza forte e fortunato sopravvive. Il nostro è un Paese in cui le prestazioni assistenziali sono spesso insufficienti, inopportune, quadri clinici e sociali che spesso risentono delle tortuose articolazioni dell'elefantiasi burocratica, diventando così scenari apocalittici. Sì, abbiamo l'apocalisse a pochi passi da casa, nel vicinato, sul nostro pianerottolo. I sindaci, gli assessori al *welfare*, i servizi sociali dei Comuni (e vi parla chi per ben dieci anni ha svolto il ruolo di capo dell'amministrazione municipale di una cittadina del Sud, Noci, in provincia di Bari) si ritrovano soli, in prima linea e diventa tutto difficile da gestire. Mettiamoci, quindi, nei panni di chi non può contare sulla benedizione di una salute intatta. Nel 2015 l'età media in Italia si è ridimensionata notevolmente. Non cresce più. Una inaspettata inversione di tendenza, una battuta d'arresto premonitrice. Ciò è conseguenza delle politiche di *welfare* funestate dalla crisi, da manovre governative di risparmio lineare e non qualitativo. finalmente è il primo disegno di legge importante sulla disabilità dal 2009, quando la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità venne ratificata. Con questo provvedimento, forse, stiamo andando nella direzione giusta, forse riusciremo a introdurre un cambiamento, un segno e un sogno di civiltà per migliaia di persone, uomini e donne. Il testo trasmessoci dalla Camera è stato notevolmente modificato e, come era intenzione, migliorato. Checché se ne dica del bicameralismo, le duplici letture consentono oggi di migliorare un testo di legge. Domani, con la pasticciata riforma costituzionale, ciò non sarà consentito. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Quindi, allorché le responsabilità piene pervadono l'azione legislativa, Camera e Senato mirano alla qualità, inseguendo il bene comune. Uno degli aspetti più "caldi" della disciplina è costituito dal *trust* e proprio su questo punto vorrei soffermarmi, perché quando parliamo di *trust* per il "dopo di noi" intendiamo un vero e proprio programma di vita. Pensiamo alle situazioni dei genitori che vogliono assicurare ai propri figli, bisognosi di particolare assistenza, un futuro il più possibile simile al presente; la maggiore diffusione dello strumento del *trust* è le cornice giuridica entro la quale i genitori rappresentano quel che dovrà avvenire da quando essi non saranno più direttamente responsabili. Ambizione legittima, genitorialità consapevole. Il *trust* è un istituto mediante il quale un soggetto disponente trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il *trustee*. Quest'ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno specifico scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell'atto istitutivo. Leggiamo in antiche carte carte notarili, che, in passato, tale disposizione veniva nominata "beneficio" e consisteva quasi in un legato. Ad esempio, ma solo per avere un'idea di quanto vado affermando, nella storia ecclesiastica delle nostre comunità di provincia, il beneficio consisteva nel godimento di sante messe di suffragio al decesso del munifico benefattore. Oggi il *trust* costituisce uno strumento flessibile, costruito su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti, per questo si inserisce nel quadro delle misure utili ad accompagnare e a proteggere le persone con disabilità nella vita quotidiana. Queste misure, a cui il *trust* può costituire non solo un'alternativa ma un aiuto complementare, sono l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Dobbiamo tenere presente che il *trust* è un istituto di origine anglosassone, la cui legittimazione, nel nostro Paese deriva dalla dalla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Con il recepimento l'Italia si impegnò a riconoscere gli effetti dei *trust* che posseggono le caratteristiche di cui all'articolo 2 della stessa Convenzione, senza però avere una disciplina interna generale della materia. Ciò ha portato allo svilupparsi di orientamenti contrastanti in dottrina, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione del *trust* interno, cioè quello in cui l'unico elemento d'internazionalità della fattispecie è rappresentato dalla legge regolatrice. Nemmeno l'introduzione dell'articolo 2645-*ter* del codice civile, che all'inizio venne salutata come la «risposta» dell'ordinamento italiano al *trust* di origine anglosassone, colmò tale lacuna. Tanto è vero che poco dopo l'entrata in vigore della norma la giurisprudenza si pronunciò nel senso che questa non avrebbe introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di negozio di destinazione, ma soltanto «un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico». Per questi motivi il "dopo di noi" dal punto di vista del *trust* è un provvedimento assolutamente innovativo, poiché costituisce a tutti gli effetti l'inedita occasione in cui viene introdotta nel nostro ordinamento una disciplina del *trust*,

che hanno seguito attivamente, che hanno vissuto sulle proprie spalle l'esperienza di una famiglia con un figlio disabile. So anche, e penso di condividere il pensiero della collega Bignami, che forse è una disgrazia, ma è anche un'opportunità e un evento che sa far crescere le famiglie; chi ha infatti una realtà come questa, ha la possibilità di affrontare sicuramente un'esperienza difficile e dura, ma estremamente accrescitiva. È da queste famiglie che noi dobbiamo trarre esempio e ispirazione anche nel momento in cui andiamo a varare questi provvedimenti. È una legge in realtà attesa da tempo. Sono provvedimenti normativi dei quali è richiesta l'emanazione e che si dovevano fare prima; prima e forse anche meglio. Ci sono già delle iniziative a livello territoriale per cercare di dare una risposta alle famiglie. Ci sono delle iniziative che però sono state lasciate quasi da sole. Nel territorio dal quale provengo, Vicenza, in particolare proprio dalla valle in cui vivo, sono partiti con un progetto pilota per cercare di creare una struttura abitativa,

grande anche sotto il profilo squisitamente economico, ma che diventa assolutamente necessario. Certo è che a fronte di tutta questa attesa ci troviamo una norma che probabilmente non sa dare una risposta all'angoscia di queste famiglie, dei genitori, di chi accudisce una persona disabile in merito a quello che sarà il futuro, che non è solo il futuro della malattia e dell'esito, ma il futuro di quello che può accadere dopo che viene a mancare il sostegno alla persona disabile. È questo il problema; c'è una difficoltà che si unisce all'angoscia e alla preoccupazione per il futuro. Una difficoltà nel crescere e curare un figlio, un familiare che è affetto da questa disabilità, pur ricordando quello che abbiamo detto circa la grande forza, l'enorme forza

prima del noi c'è la famiglia, "dopo di noi" devono esserci anche le istituzioni. È questa una grave mancanza e una grave difficoltà in cui si trova la nostra società. Per dare effettivamente un supporto serio a questa norma e a tutte le previsioni che vogliamo inventare sui *trust* o sulle donazioni, quello che dobbiamo ricordare

ciò deve essere fatto con degli interventi mirati, che purtroppo sono venuti a mancare negli ultimi anni, perché le politiche della famiglia non esistono, le politiche a supporto della famiglia mancano. Siamo arrivati addirittura a dei provvedimenti che hanno messo in discussione la famiglia in sé. Ricordate l'ampio dibattito che abbiamo avuto proprio sul tema delle unioni civili? A prescindere dall'opinione su quel provvedimento, quanto meno si è parlato di famiglia, per una volta. In qualche termine, si sono aperti dei salotti e dei confronti, dove si è detto che cos'è la famiglia.

perché, se non c'è un effettivo supporto, anche economico, a queste famiglie, non si riesce a supportare questo tipo di episodi. Possiamo parlare mille volte del "dopo di noi", possiamo dire mille volte che ci devono essere delle strutture; però alla fine la famiglia è lasciata fuori. è lasciata fuori. È ovvio quello che si vuole credere e pensare, ma la prioritaria strategia che si dovrebbe seguire è quella che dovrebbe permettere il mantenimento delle persone disabili nel nucleo della famiglia. Il problema è poi quando viene a mancare la famiglia.

è strutturata in maniera quasi mononucleare. Ormai ci si trova con una famiglia composta dal papà, dalla mamma e dai figli, mentre un tempo esistevano delle strutture sociali diverse, dove la famiglia era ampliata

Oggi invece ci troviamo con famiglie estremamente sole, dove in realtà forse il senso della famiglia viene anche a mancare, perché non c'è nemmeno più il tempo di stare assieme, perché ormai si lavora tutti: lavora il padre e lavora la madre, si lavora fino ad età avanzate, si continua a lavorare e non c'è più il tempo di stare a casa per accudire e per far crescere i figli, per seguire gli anziani e per seguire, accudire e curare anche i disabili. Quindi in questo sistema di famiglia, finché non affrontiamo il problema della famiglia, è difficile che possiamo parlare anche del problema del "dopo di noi". Il problema del "dopo di noi" è complesso, ma sicuramente quanto meno un tassello lo si comincia a mettere; si deve comunque cercare di affrontarlo raccogliendo e condividendo gli spunti che sono stati dati in quest'Aula da molti colleghi, che si sono interessati direttamente alla problematica. Per cui auspichiamo e invitiamo il Governo e la maggioranza a valutare, anche in sede emendativa, le proposte che verranno presentate ed illustrate,

Dobbiamo dare degli interventi normativi seri, che non siano solo dei belletti, ma che devono essere estremamente incisivi per dare effettivamente un supporto alla nostra società, a queste problematiche e a queste situazioni.

che oggi in Italia, come è stato ricordato, è fornito per il 68,2 per cento da genitori e, quando loro non ci sono più, da sorelle, fratelli e altri familiari. Il prendersi cura è un concetto a noi molto caro, che va oltre e comprende quello essenziale e irrinunciabile di assistenza. La legge sul "dopo di noi" vuole prendersi cura dei cittadini con disabilità, immaginando un percorso che prepara questo "dopo", una serie di servizi che si dovrebbero integrare progressivamente nel contesto familiare, in maniera da poter affrontare al meglio i cambiamenti definitivi che si impongono quanto un genitore o un altro familiare, che fino a quel momento avevano assicurato la cura, vengono meno. Quando si parla di disabilità non si parla un fenomeno marginale, non è così. Questa misura interessa il 15 per cento delle famiglie italiane. Sono disabili circa 3 milioni di cittadine e di cittadini, circa il 5 per cento della popolazione, un numero che supera quello degli abitanti di una città come Roma. Siamo consapevoli che per chi è disabile il sostegno familiare rappresenta da sempre la più efficace e completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali e ai problemi dell'integrazione sociale; se più dei due terzi dell'assistenza ricevuta dai disabili è fornita da parenti più o meno stretti, che dedicano il loro tempo, le loro energie e le loro risorse alla cura del congiunto non autosufficiente, questo è purtroppo dovuto anche alla solitudine di fronte all'handicap con la quale ancora fanno i conti troppe famiglie. Come abbiamo sentito da alcuni colleghi (ho anche avuto modo di incontrare alcuni rappresentanti di queste associazioni), il tema della solitudine

iniziare con alcune note positive. Il suo impianto è positivo nella misura in cui punta a mettere al centro la costruzione dell'autonomia di chi è disabile come prima risposta alla preoccupazione del "dopo", costruendo un'alleanza preziosa tra relazione degli affetti e relazione professionale di cura. Finalmente si parla di disabilità e lo di fa attenzionando anche chi si prende cura è infatti la famiglia il vero oggetto della legge, o almeno lo dovrebbe essere. È anche necessario immedesimarsi nella frustrazione del figlio disabile che percepisce tutto il peso dei genitori preoccupati di cosa succederà quando loro non ci saranno più. più. Il disegno di legge introduce quindi un percorso strutturato che inizia nel "durante noi", ma poi continua con la necessaria gradualità finalizzata a garantire una esistenza adulta (adultità) dei figli disabili.

piuttosto che cosa effettivamente c'è. Chiaramente una delle perplessità che questo testo ha suscitato in tante associazioni di famiglie di disabili e di genitori

Signora Presidente, mi chiedo e chiedo ai colleghi se è stato fatto un esercizio di rassegna nel cercare di capire cosa in questi sedici anni non ha funzionato e quali sono le radici profonde delle sensazioni di isolamento che le persone e le famiglie con cittadini disabili hanno percepito e stanno percependo. Dobbiamo anche interrogarci se la legge effettivamente risponda a queste necessità. necessità. Va bene il *trust* per semplificare le procedure a chi ha la possibilità di impiegare i propri beni nel percorso "dopo di noi". Vanno bene anche gli sgravi ai premi dell'assicurazione, ma chiediamoci se queste misure coinvolgono tutti

anche a chi non ha dei beni da impiegare in un *trust*? Un altro aspetto interessante è quello di rimarcare la permanenza presso la propria abitazione, quando questo è possibile. Bisognerebbe indicare tra gli interventi finanziabili da questo fondo anche quelli finalizzati a mantenere la proprio abitazione o o un'abitazione che sia familiare per il cittadino cui gli interventi sono dedicati. Signora Presidente, un aspetto molto interessante lo si ritrova nell'articolo 8, laddove si discute della relazione alle Camere.

ma, così com'è scritto questo articolo, sembra che il *focus* sia soltanto sull'aspetto economico. Si dice, ad esempio, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9 (quindi risorse economiche). Ci si affretta anche a dire, sempre nell'articolo 8, che la relazione illustra l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni. trovo estremamente riduttivo che il dibattito sul monitoraggio debba avvenire sulle minori entrate. Mi sembra veramente poco edificante.

quello che c'è, che potrebbe andare bene, ma per fare in modo che il percorso "dopo di noi" diventi un percorso di cittadinanza garantito a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro condizione iniziale. Se noi riusciremo a fare questo, riusciremo a fare di questo provvedimento davvero una buona legge.

intervengo molto brevemente. C'è una questione che ho sollevato con un'apposita interrogazione

per una ragione molto semplice. Ormai è già in vigore e si sta applicando, da parte di Poste italiane, la modalità di notifica a giorni alterni (un giorno sì ed uno no) della posta ad alcuni cittadini italiani a differenza di altri: lo dico perché nelle zone marginali del Paese è già in funzione questa modalità. modalità. L'interrogazione presentata ha esattamente l'obiettivo di sapere se l'universalità del sistema che Poste italiane deve garantire possa conoscere cittadini di serie A e cittadini di serie B, se sia immaginabile, visto il tipo di concessione che hanno le Poste italiane, un trattamento diversificato a seconda di dove abiti il cittadino, di dove risiede: